nella serata del 25 luglio 2020, in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

della Repubblica presso il Tribunale di Palermo il 31 gennaio 2020». La relazione è stata stampata e distribuita.

del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

la proposta di non autorizzare il processo, come lei ricordava, è stata approvata a maggioranza dalla Giunta. ai fatti, con comunicazione del novembre 2019 il procuratore della Repubblica di Palermo, sulla scorta delle notizie acquisite dalla procura della Repubblica di Agrigento, ha chiesto al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Palermo di procedere a indagini nei confronti del senatore Matteo Salvini, allora Ministro dell'interno, in relazione a diverse ipotesi di reato inerenti a fatti verificatesi nell'agosto 2019, riguardanti immigrati di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019 a bordo della nave Open Arms. In data 1° agosto 2019, a seguito di informazioni ricevute via *e-mail*, la nave Open Arms, battente bandiera spagnola, noleggiata dall'organizzazione non governativa Proactiva Proactiva Open Arms, effettuava, in un'area di soccorso di competenza libica, il salvataggio di 55 persone che si trovavano a bordo di un natante, dandone notizia alle autorità libiche, italiane e maltesi. In pari data, il 1° agosto, l'allora Ministro dell'interno, sottolineo - con i Ministri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, emetteva un decreto, disponendo il divieto di ingresso, transito e sosta Il 2 agosto la stessa nave effettuava un ulteriore salvataggio di 69 persone in area di competenza maltese. Di questi eventi venivano informate le varie autorità e Malta contestava la propria competenza (cosa che, com'è noto, fa spesso anche quando essa è evidente). Dopo aver

2019, Open Arms ha eseguito, con il coordinamento delle autorità maltesi, un ulteriore salvataggio di 39 immigrati. Rivolte le varie richieste, Malta si rendeva disponibile soltanto allo sbarco dei 39 immigrati salvati in quest'ulteriore operazione nelle proprie acque di competenza e contestava la possibilità di accogliere gli altri che, intanto, erano a bordo già da vari giorni.

amministrativo. Il 15 agosto, dopo un'ulteriore richiesta di POS, la nave si è avvicinata a Lampedusa, dove è stata autorizzata a collocarsi per mettersi al riparo, visto che le condizioni meteo-marine erano peggiorate e quindi vi era una necessità di salvaguardia. Vi sono poi state ulteriori iniziative di sbarco di persone che, per ragioni sanitarie, sono state fatte scendere dalla nave, con l'intervento della Capitaneria di porto italiana e della Guardia di finanza. Il 14 agosto il presidente del Consiglio Conte inviava all'allora ministro dell'interno Salvini una lettera, che è agli atti della Commissione e che anche i colleghi avranno potuto consultare, in cui lo invitava «ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare assistenza e tutela ai minori presenti sull'imbarcazione». Il giorno successivo, il 15 agosto, l'allora ministro dell'interno Salvini rispondeva con una lettera, dicendo che, avendo la nave bandiera spagnola, doveva essere quel Paese ad averne la giurisdizione, quindi anche la competenza, per quanto riguardava i minori e la tutela dei loro diritti umani. umani. Salvini faceva presente che c'erano anche adulti che accompagnavano i minori. Il 16 agosto, dopo un'ulteriore evacuazione per ragioni sanitarie e la notifica di un atto extragiudiziale di diffida, con cui i legali della Open Arms chiedevano a vari Ministri di autorizzare l'ingresso della nave nel porto, il Presidente del Consiglio, replicando alla risposta che aveva ricevuto dal ministro Salvini, evidenziava la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo. Richiamo l'attenzione dei colleghi, perché è su questi fatti che dobbiamo votare, non su una discussione astrattamente politica, che potrebbe svolgersi in altre sedi e in altri luoghi: il Presidente del Consiglio indicava la necessità di far sbarcare i minori, con una lettera. Il ministro Salvini rispondeva a tale invito il 17 agosto (quindi le risposte erano immediate, da un giorno all'altro, ovviamente, considerate la delicatezza e l'attualità della vicenda), assicurando che, nonostante non condividesse la lettura della normativa proposta dal presidente Conte, avrebbe

Il Ministro quindi si uniformava alla direttiva del Presidente del Consiglio, riconoscendone ovviamente l'autorità gerarchica superiore. Non mi dilungo sulle norme della Costituzione e sul ruolo del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei ministri; anzi, a maggior ragione, non condividendo, dimostrava di eseguire una direttiva e pertanto il coinvolgimento del Governo nelle massime gerarchie è evidente e palese. Già qui mi potrei fermare, colleghi, nella mia relazione sui fatti, perché di questo ci occupiamo oggi: il resto fa parte del quotidiano dibattito politico, né citerò nella mia relazione fatti di attualità che ho letto anch'io sui giornali e che tuttavia non rientrano nei miei compiti e nelle mie funzioni di relatore, rispetto alle polemiche sulle intercettazioni, che non sono state, non possono e non devono essere oggetto non devono essere oggetto della valutazione della Giunta, ma fanno parte della discussione politica. Il 18 agosto, su disposizione della prefettura di Agrigento e dietro comunicazione dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno, i 27 minori non accompagnati venivano fatti sbarcare a Lampedusa. Nel frattempo, le autorità spagnole autorizzavano lo sbarco della nave

I minori erano quindi stati fatti sbarcare, perché il Ministro dell'interno aveva accettato ovviamente l'indicazione e la disposizione del Presidente del Consiglio. Successivamente, il 20 agosto,

dopo che i minori erano stati fatti scendere, in ottemperanza a un indirizzo di Governo. Si discute sulla natura di quest'atto. Il collegio per i reati ministeriali ha escluso quella di atto politico delle condotte ascritte e vi ha riconosciuto invece invece un reato ministeriale, chiedendo al Senato l'autorizzazione a procedere, contro la quale la Giunta si è espressa. Quindi, la relazione che sto qui rappresentando è espressione dell'orientamento della Giunta, contraria all'autorizzazione Vi risparmio lunghe considerazioni in termini di diritto, che potrete trovare nel testo della relazione, che vi prego di approfondire, per collocare bene, in termini giuridici, la decisione e il voto che Nel caso di specie, va sottolineato che il tribunale dei Ministri, valutata la riconducibilità della condotta del ministro Salvini a reati, astrattamente ipotizzati, di sequestro di persona e di rifiuto di atti d'ufficio, ha ravvisato la natura ministeriale dei reati stessi e ha proceduto alla formulazione dei capi d'imputazione, sui quali il Senato sarà chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti, previsti dall'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 per il rilascio dell'autorizzazione a procedere. Non c'entrano niente l'articolo 68 o altri aspetti Grazie a tutti

C'è tutta una giurisprudenza che ci ha aiutato nell'esame delle vicende (questa è la terza e ognuna ha una sua specificità), però le materie, le fonti del diritto, i precedenti e le sentenze del Consiglio di Stato sono alla base delle motivazioni che abbiamo già rappresentato in altri casi all'Assemblea e che negli atti sono specificate, ragion per cui non mi ci soffermo, non perché non siano importanti, ma perché sarebbe faticoso seguire nel dettaglio le innumerevoli siamo quindi di fronte a una scriminante ai sensi del codice penale, che consente a chiunque di impedire un fatto dannoso; qui siamo nel fatto specifico di un'azione di Governo. Abbiamo visto in alcuni casi fare anche confusione con l'articolo 51 del codice penale, ma qui siamo in un'altra

se vi fosse traccia della *moral suasion* dell'azione del Presidente del Consiglio. Anche per esperienza personale, so che, quando si riunisce il Governo, il Presidente del Consiglio dà indirizzi, corregge posizioni e invita alla riflessione

Ovviamente, non possiamo chiedere alla Presidenza del Consiglio prove di quest'azione, che è di indirizzo e spesso non lascia tracce formali scritte. Nella relazione è citata una sentenza della Corte costituzionale

alle nomine di competenza delle alte sfere dello Stato: non sempre troverete un verbale, ma certamente ci sono un confronto e una discussione. La sentenza che riguarda il Presidente della Repubblica

con le conseguenze politiche del caso. Egli ha ottemperato a quella direttiva. Peraltro, si deduce che il Presidente del Consiglio dei ministri dell'epoca, se avesse voluto disporre lo sbarco di tutti,

che evidentemente non ha ritenuto di emanare; in termini di *moral suasion,* di attività di indirizzo e di coordinamento del Governo, egli

- che dobbiamo occuparci. La discussione puramente politica riguarda altri ambiti e, come ricordo nella relazione, si possono presentare interrogazioni, mozioni di sfiducia

l'uniformità dell'azione del Ministro dell'interno alle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri; lo sbarco concesso in Spagna, con il POS ad Algeciras; il non gradimento della località lontana; lo sbarco più vicino nelle Baleari; la disponibilità della Capitaneria di porto ad affiancare l'Open Arms con una nave italiana, per rendere meno disagevole la trasferta, che comunque era affrontabile (parliamo sempre di un'area mediterranea limitata); tutto questo, insomma, ci ha portato a ritenere che si sia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. All'epoca l'interesse pubblico consisteva nella regolamentazione più rigorosa della gestione dei flussi migratori per disincentivare il traffico degli immigrati. Sappiamo che dietro queste attività - se ne discute anche in questi giorni - ve ne sono altre criminali, che, in Libia e altrove, traggono profitto illecito dalla loro gestione.

il 13 giugno 2018) il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e le massime autorità della sicurezza hanno rilevato la possibilità di infiltrazioni terroristiche nel traffico dei clandestini. Qualcuno dirà che il Ministro sapeva quali erano, ma non

che può utilizzare il fenomeno migratorio, non perché gli immigrati che giungono siano tutti i terroristi (nessuno lo può pensare), ma perché una situazione di disordine e caos può avvantaggiare o favorire chi possa infiltrare in Italia e in Europa persone che vengano qui non in cerca di pane e lavoro, ma con altri scopi. Questo pericolo è stato evidenziato nel corso degli anni da parte delle massime autorità della sicurezza, con relazioni e rapporti che forse neanche noi leggiamo con attenzione. Come parlamentari

coperte da segreto, ma di carattere generale. Anche in questi giorni mi è capitato di leggere sui giornali l'allarme dei servizi di sicurezza, perché sulle coste della Libia migliaia di persone con rischio di infiltrazione sono pronte a varcare il Mediterraneo. il Ministro dell'interno ha agito sulla base di questi indirizzi di Governo e anche nel perseguimento di quest'interesse pubblico. La parola «perseguimento» vuol dire che l'azione del Governo persegue quell'obiettivo, non ha la certezza di raggiungerlo. Per quanto riguarda gli atti,

ovviamente, mi chiedevo se fossero gli stessi della procura che poi hanno espresso orientamenti diversi, ma su questo forse sarà il dibattito a offrire temi di riflessione.

che ha approvato la mia proposta, il ministro Salvini ha perseguito un interesse pubblico preminente inerente all'azione di Governo, costituito dalla gestione dei flussi migratori, anche al fine di prevenire (ma questo è un fatto accessorio) una minaccia terroristica emersa in sede di Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica dal 2018 (ma credo anche in altre occasioni e sicuramente in passato). Sul piano politico, come ho già detto, ognuno può esprimere giudizi, mozioni e sfiducie, ma è un'altra cosa: in questo caso, siamo su un piano di diritto, sull'applicazione della legge del 1989 e sulla valutazione dell'azione di un Ministro e - lo lo ribadisco ancora una volta - di un'azione di Governo, ossia il decreto interministeriale contro l'arrivo della nave e le direttive epistolari, meditate e formalizzate del Presidente del Consiglio. Non stiamo parlando di telefonate, intercettate o raccolte, ma di atti formali, che sono stati anche eseguiti, pur nella divergenza di opinioni, e ciò dimostra proprio che, a un certo punto, è stata la Presidenza del Consiglio ad aver assunto la gestione di alcune scelte e ad aver imposto l'applicazione di quelle che ha ritenuto di indicare, mentre di altre evidentemente non ha ritenuto di avvalersi. Questo è il fatto, colleghi. Siccome siamo parlamentari avveduti ed informati e poiché molti, anche in quest'Aula, hanno ricoperto responsabilità di Governo a vari livelli, è conosciuta la prassi della gestione delle vicende, anche di quelle complesse, in termini di fatto e di diritto. È per questa ragione, quindi, che la Giunta

sui quali ci siamo misurati; la vicenda si è protratta anche più del necessario, perché c'è stata tutta la vicenda del rallentamento dell'attività giudiziaria del Paese; anzi, devo dire

approvare la proposta della Giunta per il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere, attesa la sussistenza, nel caso di specie, dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. Certamente non mi sfugge la rilevanza politica delle cose che discutiamo, ma ci troviamo anche in una sede che deve muoversi in base ai fatti, alle leggi, alle norme e alle prerogative che riguardano l'azione di Governo in termini astratti ed assoluti. Oggi l'interessato non svolge funzioni di Governo, ma la questione delle azioni di Governo riguarda l'istituzione nella sua complessità, nelle decisioni che deve assumere:

ampia e non cesserà mai, come è normale che sia. Su questo fatto gli elementi, a mio avviso, sono molto chiari, la Giunta ha avuto modo di discutere e anche di meditarli, perché sono rimasti ai nostri atti più del necessario, ma con una rapidità maggiore di altri livelli di giustizia, e quindi invito i colleghi ad approvare questa proposta che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'allora ministro Matteo Salvini.

per il modo in cui in tre diverse occasioni ha esercitato i poteri del Ministro dell'interno per impedire l'attracco di imbarcazioni che avevano prestato soccorso in mare e lo sbarco dei naufraghi ed è la terza volta che mi confronto, proprio a partire dalla Costituzione, con il relatore Gasparri. Per la terza volta, intervengo per ricordare a questa Assemblea qual è il compito che ci assegnano la Costituzione e la legge in questo passaggio istituzionale e soprattutto per ricordare quello che non è il nostro compito e cioè quali sono i limiti dell'esercizio del nostro potere. Partiamo da quello che non dobbiamo e non possiamo fare. In primo luogo, oggi non siamo un tribunale che deve decidere se, rispetto alle accuse, il senatore Salvini sia colpevole o innocente, se altri con lui siano responsabili dei reati che vengono loro contestati, ovvero se il giudizio disposto nei suoi confronti abbia correttamente valutato gli elementi emersi nel corso dell'indagine. non siamo chiamati né a giudicare la decisione del tribunale dei Ministri, né ad anticipare la decisione che prenderà il tribunale ordinario se il Senato consentirà il processo. In secondo luogo, in questa sede credo che non dobbiamo discutere le idee del senatore Salvini sull'immigrazione e la loro relazione con la sua condotta nel caso Open Arms come nei precedenti. Da oltre un anno aspetto il momento, che questa maggioranza continua a rinviare, in cui il Parlamento potrà discutere della modifica dei cosiddetti decreti sicurezza e della riforma della legge sull'immigrazione. non questa è la sede in cui discutere le idee, le iniziative politiche e le responsabilità del senatore Salvini.

che le norme dei decreti sicurezza ovviamente non hanno affatto cancellato. L'appello allo Stato di diritto e alla garanzia dei diritti dei cittadini, e degli imputati in primo luogo, deve essere corrisposto da ciascuno rimanendo nell'alveo del proprio potere e della propria funzione. Io non voglio e voi non potete né fare gli accusatori, né i difensori, né i giudici del senatore Salvini. Veniamo invece al nostro compito, lo ripeto: ai limiti del nostro potere. Noi dobbiamo valutare se le condotte di cui la magistratura contesta la rilevanza penale fossero finalizzate a tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero a perseguire un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. La Giunta delle immunità ha ravvisato la sussistenza di questa seconda scriminante ritenendo che il senatore Salvini abbia agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Al contrario, io ritengo che l'ex ministro Salvini abbia giustificato la propria condotta per finalità genericamente politiche, per esempio la difesa dell'interesse nazionale, di cui non è affatto scontata la coincidenza con l'interesse pubblico che infatti non è stato qualificato e di cui non è stata motivata la preminenza rispetto ad altri interessi e diritti in gioco sacrificati in quella circostanza. circostanza. La mancata qualificazione dell'interesse pubblico e di motivazione della sua preminenza è già più che sufficiente per giustificare il voto contrario al diniego all'autorizzazione perché, ripeto, come dice anche la sentenza della Corte, perché possa essere negata l'autorizzazione a procedere si deve motivare - dico bene: non affermare, ma, dice la Corte, si deve motivare - che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante. La motivazione non può essere meramente politica ma deve indicare quale sia l'interesse dello Stato. la possibilità che ci fossero terroristi a bordo. Non è così e non è così per legge, perché il rischio deve essere provato, immediato, contestuale e non previsto: previsto: per rappresentare una causa di giustificazione della condotta del Ministro avrebbero dovuto essere minacce concrete.

i motivi di sicurezza nazionale che possono giustificare la violazione della legge devono comportare reale e attuale pericolo all'integrità dello Stato, alla vita e all'incolumità delle persone, ai diritti costituzionali, cioè veri e propri stati di necessità che francamente non vedo. Quindi io penso, per queste ragioni, proprio perché non faccio il giudice, che il collega Salvini avrà, come tutti i cittadini italiani, tutte le possibilità di difendersi nel processo. Farà in quella sede le chiamate di correo o non le farà, dipende dalla strategia difensiva. il processo durerà a lungo, ma durano a lungo anche per milioni di cittadini italiani, troppo a lungo e per questo, per la terza volta, io voterò contro la proposta di negare l'autorizzazione al giudizio nei confronti del senatore Salvini. Lei, senatore Salvini, avrà un'ottima difesa, ne sono convinta.

Lei stesso ha detto: processatemi subito, perché così processate il popolo italiano. Insomma, come megalomania non è male. Senatore Salvini, lei non è il popolo italiano, lei oggi, in questa sede, è un senatore che, a mio avviso, deve rispondere dell'esercizio delle sue funzioni da Ministro e ne avrà tutte le possibilità. Non siamo noi e non deve essere il Senato lo scudo dal processo. Vi sia semmai un invito a tutti quanti, anche quando sono Ministri, ad esercitare le proprie funzioni nell'ambito e nel limite della Costituzione e delle norme vigenti.

che peraltro alcuni non attribuiscono neanche a lui, dopo un terribile fatto in Francia. Egli disse: «È peggio di un crimine. È un errore». Credo che nella vicenda della gestione della politica migratoria del Paese dal 2018 al 2019, con il cosiddetto Governo giallo-verde, prima ancora di discutere se vi siano stati crimini, cosa che non spetta a noi, come ha ricordato la collega Bonino molto correttamente qualche istante fa, vi debba essere una chiara e precisa distinzione tra chi crede che sia stato un errore e chi crede che non sia stato un errore. Noi non abbiamo cambiato idea su questo fatto: lo dico ai colleghi del MoVimento 5 Stelle. Noi abbiamo sempre pensato che quella gestione di politica migratoria fosse un errore

a quella parte degli intellettuali della sinistra che hanno inteso stabilire una connessione tra Governi profondamente diversi, tra persone politiche profondamente diverse, unite forse soltanto dal nome di battesimo e che hanno sostenuto in questi anni che noi eravamo la brutta copia della destra, quando andavamo a salvare non soltanto le persone in mare, ma anche - lo sa l'*ex* ministra Pinotti - a raccogliere in mare, con la Marina militare, i cadaveri dei migranti deceduti nel corso della traversata. Noi eravamo questo: una cosa diversa da voi. Noi eravamo quelli che mettevano i soldi nella cooperazione internazionale, perché dire «aiutiamoli a casa loro» per noi era un principio giusto, da realizzare concretamente, aumentando i fondi alla cooperazione internazionale, cosa che questa parte dell'emiciclo ha fatto, quando ha governato, e che quella parte dell'emiciclo non ha fatto, quando ha governato. Noi eravamo quelli che, contro l'opinione dei più, volevano lo *ius culturae* e che pensavano che, se si volesse davvero combattere il disinteresse dell'Europa, occorresse almeno andare alle riunioni in Europa, cui il ministro Salvini ha partecipato raramente.

passate esperienze professionali e politiche, che è il rapporto tra la magistratura e la politica. Questi sono i due punti in più. Chiarito che politicamente noi siamo da una parte e voi dall'altra e che qualcuno ha cambiato idea nel corso degli anni - meno male!

né se Salvini in questo reato fosse in qualche misura accompagnato da altri membri del Governo. A questa domanda deve dare una risposta la magistratura. Noi dobbiamo dire se vi era un interesse costituzionalmente tutelato e/o un preminente interesse pubblico nella scelta del senatore Salvini di non far sbarcare i migranti, scelta che il Presidente del Consiglio avalla, almeno nella parte in cui non fa riferimento ai maggiorenni nella sua lettera che ricordava il presidente Gasparri. Questa è la domanda io rispondo dicendo che per me l'interesse costituzionale tutelato o il preminente interesse pubblico in questa vicenda non ci sono, come non c'erano sulle precedenti due richieste di autorizzazione a procedere. Io non posso dire che esista un interesse pubblico preminente nel tenere un barcone lontano dalle coste italiane. Posso discutere delle scelte politiche e ritengo questa valutazione una scelta finalizzata a strumentalizzare il consenso. Tu non blocchi l'immigrazione tenendo un barcone al largo, tu aumenti i *follower* su Facebook. È la visione È la visione populista dell'immigrazione, perché se vuoi bloccare l'immigrazione devi gestire a monte i processi, devi andare a fare un grande investimento in Africa, devi avere una visione europea, devi partecipare alle riunioni europee, devi fare esattamente il contrario di quello che il primo Governo Conte ha fatto. Il punto politico è che di fronte a questo passaggio le considerazioni che vengono espresse dai colleghi della Lega e in modo più istituzionalmente corretto dal presidente della Giunta delle sono assolutamente corrette nella parte in cui dicono che vi è una responsabilità condivisa con il Governo. Qui nessuno può negare questo fatto; non lo può negare la sinistra, non lo può negare la destra, ma non è l'elemento del contendere. Anzi, dico con molta franchezza, noi che abbiamo votato a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini e che ci accingiamo a votare nuovamente a favore, diciamo in quest'Aula che se vi fosse una richiesta di autorizzazione a procedere non già contro l'ex Ministro dell'interno, senatore, ma contro l'ex Ministro dei trasporti, anch'egli coinvolto nella gestione dei porti, noi voteremmo allo stesso modo per l'autorizzazione a procedere. Se infatti non c'è l'interesse pubblico preminente per il senatore Salvini, non c'è neanche per il senatore Toninelli.

che vi siano delle *chat* di magistrati in cui si dica che un parlamentare, in questo caso un mio avversario politico, ma un parlamentare che deve godere del rispetto di questa Aula *(Applausi)*, debba essere attaccato, a prescindere, anche se ha ragione.

il punto politico è che la politica rispetta l'articolo 96 della Costituzione, visto che vi sciacquate la bocca della Costituzione, in pausa pranzo fate almeno uno sforzo per leggerla. È una dotta citazione

Io non ho fretta ed è evidente che chi in queste vicende non riesce a passare dal populismo alla politica, non riesce cioè a capire che, quando si è in Parlamento e si volta su un'autorizzazione a procedere, non si vota su un *tweet*, ma su un articolo della Costituzione che va quantomeno letto, dimostra di vivere oggi quella legge del contrappasso per cui quel populismo che era la ragione per la quale si bloccavano i barconi oggi vi si ritorce contro. *(Commenti)*. Vengo al secondo punto. Il rapporto tra la magistratura e la politica è un rapporto nel quale abbiamo un elefante nella stanza, signor Presidente. Il 12 dicembre, intervenendo in quest'Aula, avevamo chiesto una riflessione politica matura. Allora ci fu detto di no, perché allora la questione riguardava il finanziamento alla politica per il tramite di una fondazione che veniva giudicata corrente di partito. o affrontiamo il tema del rapporto tra magistratura e politica oppure prima o poi tocca a tutti. Cerchiamo di essere chiari: se una componente articolata di un partito viene così definita, anche se è una fondazione che organizza eventi, e pertanto si applica a costoro la legge sul finanziamento illecito ai partiti, pur essendo in presenza di un fatto giuridico diverso e di una configurazione giuridica diversa, se questo accade oggi per una fondazione, quale che essa sia, domani può accadere che una srl che lavora a fianco della politica può diventare il soggetto cui viene contestato un finanziamento illecito alla politica. politica. Amici e colleghi, quello che esce dalle intercettazioni dei magistrati è stato casualmente e improvvisamente messo in naftalina da tutti i principali organi di informazione. Perché, signora Presidente? Se queste informazioni, che vengono da dei magistrati, fossero uscite da dei politici, quei politici sarebbero tutti indagati come minimo per traffico di influenze. Se ci sono degli strumenti come i *trojan* - lo dico qui in Senato, e non mi riguarda - che vengono accesi e spenti senza un criterio logico; se rimangono accesi, nonostante la diversa indicazione del magistrato inquirente, a fronte della presenza di parlamentari in una riunione - questo è un atto gravissimo, sul quale bisognerà che lei, signor Presidente, con il suo collega Presidente della Camera, prima o poi intervenga - se i *trojan* rimangono accesi quando c'è un parlamentare, se il *trojan* rimane acceso quando c'è un incontro molto privato, intimo, della persona sotto indagine e se improvvisamente il *trojan* si cancella quando si incontra qualcun altro, magari perché è un personaggio importante delle istituzioni o della magistratura, siamo in presenza di una deriva

viviamo una stagione politica complicata, in cui un magistrato serio e bravo, che si iscrive ora alla scuola di Castelpulci, rischia di non fare la stessa carriera di un altro suo collega, magari meno bravo, perché non si iscrive alla corrente giusta o magari perché non si iscrive ad alcuna corrente.

correttamente, sulla base della sentenza ma che oggi vede la propria vicenda personale profondamente rimessa in discussione da alcune intercettazioni e registrazioni di un magistrato. Siamo cioè in presenza di un fatto: il fatto è che c'è un... che non funziona. Qui ci sono due alternative. La prima è che voi pensiate di prendere il singolo atto e di ragionare su di esso; in questo caso, l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Salvini. Non c'entra niente, perché lì c'è l'articolo 96 della Costituzione. La seconda La seconda è avere il coraggio, maggioranza e opposizione insieme, di mettersi intorno a un tavolo a cominciare da settembre, signor Presidente, e di discutere del rapporto tra politica e magistratura, sapendo che da questa parte del tavolo troverete persone pronte ad ascoltarvi. Ma da questa parte della maggioranza deve essere chiaro: non domandatevi per chi suona la campana, perché una volta suona per qualcuno, una volta suona per altri, ma presto potrebbe suonare per chi non se l'aspetta. Abbiamo il coraggio di affrontare finalmente la questione del rapporto tra politica e magistratura.

dico rispettosamente al collega Renzi -mi pare tanto affermare questo, ma ci provo - di trarre le conseguenze. Dal punto di vista giuridico, secondo me,

ma per la complessità della materia, che è stata trattata - come si dice - in punta di diritto riguardo al pregresso, alle sentenze precedenti e anche nel particolare momento storico. Se andiamo a esaminare le decisioni discrezionali di Salvini, la lettera di Conte a riguardo dell'obbligo, necessità e consiglio di far sbarcare i bambini, l'aver fatto sbarcare gli ammalati,

mi domando se la quarantena disposta in queste settimane sulle navi, peraltro a costi proibitivi, non sia una forma indiretta di sequestro. Che differenza c'è? C'erano più servizi sulle navi che facevano quarantena? C'era un'area giochi o qualcosa di diverso? Ma voglio tornare alla questione essenzialmente come si può agire politicamente e come si possono tradurre le scelte politiche in atti amministrativi. In altre parole, voglio parlare della discrezionalità dell'azione politica e amministrativa, che è un tema che è stato oggetto di sentenze, sentenze, scritti e dibattiti e che non si è mai risolto perché, per sua natura, non può essere risolto in quanto in tanti casi la materia e soprattutto le decisioni si accavallano e creano delle impossibilità a dirimere. Un programma politico e la difesa di interessi collettivi diffusi, che sono giudicati preminenti da una parte politica che rappresenta una parte predominante del corpo elettorale, come possono essere tradotti, quando il confine è labile? Allora, la discrezionalità, a mio avviso, va interpretata in questo e in altri casi con alta possibilità di analogia e di interpretazione largheggiante, con prevalenza della politica come interesse collettivo degno di essere difeso. Intanto e in fondo su questa questione siamo sempre a parlare della differente concezione dell'immigrazione e di ciò che sta succedendo. Ogni tanto mi interrogo da cristiano se, essendo contrario all'immigrazione, sono nella giusta interpretazione e traduzione del magistero. Poi, mi confronto e mi consolo con quanto dicevano Wojtyla e Ratzinger - un po' meno con quanto dice il papato recente - e mi autogiustifico, come facciamo tutti oggi, che siamo tutti diventati un po' protestanti e ci confessiamo da soli. se non c'è, in fondo, una motivazione religiosa secondo la quale io, noi, un partito, una fazione, uno Stato è portato a dire che accetta tutti coloro che arrivano in Italia e ha questa tensione profonda, se è soltanto per altri motivi, allora non ci siamo. Giustifico il cristiano che interpreta in una certa maniera, un po' integralista, il concetto di immigrazione, ma per un cittadino, per un italiano, che non è obbligato a pensarla in questo modo, non posso giustificare quello che è successo e quello che succede in queste settimane. Far arrivare tutti, come sta di nuovo non è un reato contro i cittadini italiani più deboli? Perché sottrae *welfare*, c'è poco da fare: se c'è uno stanziamento di 1 milione di euro o di un 1 miliardo per il *welfare* e arrivano mille persone, è un conto, ma se ne arriva 1 milione, è un altro conto: non posso soddisfare tutti, Tutto ciò crea insicurezza. Mi dicono che è soltanto percepita. No, è insicurezza reale; sono cambiati gli stili di vita, soprattutto in certe zone del nostro Paese. Ma perché - vi dicevo - una famiglia di italiani che era emigrata dal Sud a Torino e che aveva comprato a fatica un alloggio in un condominio, in cui gli altri alloggi sono stati acquistati successivamente da immigrati (in parte, in realtà, sono stati anche occupati), oggi si trova costretta a svendere o a regalare quell'alloggio? Ma cosa ne può quella famiglia di italiani che ha lavorato una vita e la moglie è andata pure a pulire le scale di lor signori? C'è qualcosa che non quadra. Io sono dalla parte di quegli italiani deboli. all'utile che favorisce alcune cooperative, le ONG che hanno sedi negli Stati più strani ma mai in Italia: li portassero in Olanda, in Spagna o dove piace a loro o dove battono bandiera. Si rinuncia Si rinuncia ai valori fondamentali della nostra civiltà, ai nostri valori di democrazia e di società, per creare un tipo di popolo di cui non si capisce più né l'origine né la storia né il futuro. Ma, secondo voi, visto quello che hanno pubblicato i giornali (a meno che non siano fotografie false), chi arriva con il barboncino è uno che ha problemi economici e che scappa dalla guerra? C'è una falsa rappresentazione della realtà che è data anche dalla televisione e dai *media*, per cui in Africa si pensa che qui sia tutto gratis e tutto sia dovuto. Se poi arrivano con il virus, diciamo: ma no, proibiamo piuttosto gli ingressi ai turisti, come abbiamo fatto l'altro ieri, con la proroga dello stato di emergenza. Il turismo è in difficoltà, allora che facciamo? Non possono arrivare i turisti stranieri che spendono? No, quello è peccato; facciamo arrivare gli immigrati e se hanno il virus e poi scappano, pazienza, triste a chi tocca. Perché non tocca quelli che stanno al centro di Roma o che stanno in certi tipi di palazzi e frequentano certi ambienti. E questo lo dice uno di centrodestra. Questo per dire che qui il voto è essenzialmente politico, è essenzialmente politico, a seconda se si è in maggioranza con Salvini o si è in maggioranza senza Salvini; a seconda delle sensazioni.

compatta; poi, ieri sera e questa notte abbiamo visto quanto fosse compatta. Io vi dico: in questo voto siate compatti come nella serata di ieri e nella notte scorsa, e Salvini si salverà.

siamo nel solco dell'articolo 96 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1989 (articolo 9, comma 3), così come per le due fattispecie che ci hanno occupato in precedenza, il caso Diciotti e il caso Gregoretti. Vorrei soffermarmi però su un passaggio squisitamente tecnico che va ad intersecarsi con un dato politico, che è stato pur giustamente evidenziato. In data 1° agosto 2019, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emetteva un decreto con il quale disponeva «"sin da ora" il divieto di ingresso, transito e sosta della nave Open Arms "nel mare territoriale nazionale"». Ho riportato il brano testualmente. Il 14 agosto 2019 il presidente del TAR Lazio emetteva un decreto monocratico, ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, con il quale accoglieva testualmente - «nei sensi di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari monocratiche» della ricorrente ProActiva Open Arms, nell'ambito del ricorso per annullamento del sopracitato provvedimento interministeriale. il presidente del TAR Lazio, in ordine al *fumus* osservava che il ricorso non appariva «del tutto sfornito di fondamento giuridico» in relazione al vizio dedotto, mentre con riguardo al *periculum in mora* riteneva che sicuramente sussistesse, «alla luce della documentazione prodotta», «la prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza», testualmente - «tale da giustificare la concessione - nelle more della trattazione dell'istanza cautelare nei modi ordinari - della richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l'ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane (e quindi di prestare l'immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli, come del resto sembra sia già avvenuto per i casi più critici)». Appare quindi Appare quindi chiaro, *per tabulas* e senza alcuna ombra di dubbio, che la portata del decreto monocratico del presidente del TAR era circoscritta all'ingresso nelle acque territoriali, al fine di consentire assistenza sanitaria e materiale alle persone più bisognevoli. Nessun obbligo di sbarco può desumersi da tale atto giudiziario. Peraltro, ove il presidente del TAR avesse voluto ordinare lo sbarco, avrebbe sancito espressamente tale obbligo, anche in ossequio al principio metodologico generale dell'*ubi lex voluit ibi dixit, ubi noluit tacuit*, principio concepito per il legislatore e per le leggi, ma sicuramente estensibile anche agli atti giudiziari, atteso che esigenze di certezza del diritto risultano incompatibili, sia a livello di leggi, che di atti giudiziari, con profili taciti e inespressi, presupponendo al contrario statuizioni esplicite e chiare. Nella missiva del 15 agosto 2019 l'allora ministro Salvini riferiva al presidente Conte di avere dato mandato in ogni caso all'Avvocatura generale dello Stato di impugnare il menzionato decreto. Si segnala che il 19 agosto 2019 il vice capo di gabinetto del Ministero dell'interno, il prefetto Formicola, in relazione alla richiesta di assegnazione POS (Place Of Safety), chiariva come, secondo la prospettiva del Ministero, il decreto interministeriale del 1° agosto non avesse cessato di produrre i suoi effetti alla luce del provvedimento cautelare del presidente del TAR Lazio, con il quale si erano unicamente indicate misure cautelari d'urgenza, finalizzate a consentire l'ingresso del natante in acque territoriali per garantire assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli, non imponendo alle autorità italiane alcun obbligo in ordine all'assegnazione di un porto di sbarco nel territorio nazionale. Sottolineava, inoltre, che le stesse autorità italiane avevano adempiuto ai doveri di assistenza, concorrendo nell'effettuazione delle evacuazioni mediche necessarie e curando lo sbarco di 27 minori non accompagnati e presenti a bordo. Il senatore Salvini, anche nella memoria depositata in Giunta il 17 febbraio 2020, precisa che il 19 agosto 2019 il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri presentavano innanzi al TAR TAR Lazio istanza di revoca del decreto cautelare del presidente del TAR Lazio, ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo, stante l'inesistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto, nonché per essere stata sempre assicurata l'assistenza medica a tutti i migranti, come dimostrato dalle evacuazioni mediche, non potendo così la nave sostare ulteriormente in acque territoriali italiane. In pari data, quindi sempre il 19 agosto 2019, la Open Arms produceva dinanzi al TAR Lazio una memoria per contrastare la suddetta istanza di revoca, formulando richiesta di nuovo provvedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 56, comma quarto, del codice del processo amministrativo, chiedendo al presidente dello stesso TAR, previa conferma del precedente decreto, di adottare, leggo testualmente: «ad integrazione dello stesso tutte le misure necessarie per consentire lo sbarco di tutti i migranti». Appare evidente che la tesi secondo cui il decreto monocratico del presidente del avrebbe imposto lo sbarco, non solo contrasta con la lettera del provvedimento stesso, come già sottolineato, ma appare del tutto incompatibile con lo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, con quello di Open Arms, che non avrebbe mai chiesto un secondo decreto per ordinare lo sbarco, ove lo sbarco fosse già stato ordinato nel primo decreto. In altri termini, gli stessi legali di Open Arms presentarono nuova istanza di ulteriore provvedimento cautelare che ordinasse lo sbarco dei migranti, confermando in tal modo la non satisfattività del provvedimento cautelare monocratico rispetto alle pretese di quella parte processuale. Va sottolineato, inoltre, che, qualora il decreto avesse ordinato lo sbarco e fosse rimasto inadempiuto, i legali di Open Arms si sarebbero sicuramente avvalsi dell'articolo 59 del codice del processo amministrativo, il quale prevede che, «qualora i provvedimenti cautelari non siano eseguiti, in tutto o in parte, l'interessato, con istanza motivata e notificata alle altre parti, può chiedere al tribunale amministrativo regionale le opportune misure attuative». Il tribunale, in tal caso, come precisa espressamente tale disposizione, esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza. Nel caso di specie, nessuna ottemperanza ai sensi del citato articolo 59 è stata richiesta, perché non era in alcun modo stato disposto lo sbarco. Non può essere, quindi, individuata alcuna strada che consenta di ritenere che il primo decreto monocratico del presidente del TAR avesse ordinato lo sbarco. Tale assunto emerge dalla lettera del provvedimento in questione ed è altresì confermato ulteriormente dai comportamenti assunti dagli stessi legali di Open Arms rispetto a tale atto giudiziario. La suddetta incompatibilità logica della concessione del *place of safety* (POS) con il citato decreto, riconosciuta finanche dal tribunale, palesa quindi il fine politico e l'inesigibilità di un comportamento diverso, che sarebbe stato difforme dalla concertazione posta in essere. La vicenda di Open Arms è quindi pienamente ascrivibile all'esercizio della funzione di Governo per il perseguimento di obiettivi di politica migratoria, tesi a contrastare il traffico di esseri umani e a richiamare gli altri Stati membri dell'Unione europea, così come previsto dall'accordo del Consiglio d'Europa del 28 giugno 2018, ad un onere di condivisione nella gestione del fenomeno, fin dalle operazioni di ricerca e di soccorso in mare. Le azioni poste in essere dal Ministro dell'interno si erano pertanto realizzate in attuazione di un indirizzo politico del Governo, così come documentato nelle precedenti fattispecie che ci hanno occupato, a seguito anche della lettura delle memorie del Presidente del Consiglio e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dell'epoca, che confermavano questa linea di politica generale del Governo. *(Applausi).*

del senatore Salvini e del modo in cui ha esercitato la funzione ministeriale. Ho appena finito di ascoltare la relazione del collega e amico Urraro, molto interessante

è irrilevante. Noi infatti dobbiamo occuparci oggi di una questione che temporalmente si inquadra tra il 14 e il 20 agosto 2019. In questo arco temporale abbiamo una situazione politica abbastanza delineata e definita, poiché dal giorno 8 il senatore Salvini aveva, masochisticamente direi, minacciato di staccare la spina a un Governo del quale non si era reso conto di essere il *leader*; di fatto, era il *leader*. Che fosse il *leader* si vede dagli atti che furono posti in essere da quel Governo, ad esempio, come diremo, con il decreto sicurezza-*bis*. Voleva staccare la spina il giorno 8, poi però non ebbe il coraggio di andare oltre e non si dimise. Quando uno fa le cose in questo modo, dal punto di vista umano, politico e sociale, chiaramente poi ne paga...

Era la seguente. Open Arms aveva effettuato alcune operazioni di soccorso in mare. Era stato emanato, ai sensi del decreto sicurezza-*bis*, un decreto interdittivo, come ha ben detto il collega Urraro, che impediva alla nave di entrare nelle acque territoriali e di effettuare lo sbarco dei naufraghi (si parla infatti di persone raccolte in mare in procinto di annegare). Questa situazione, però, a un certo punto era stata affrontata da Open Arms, che aveva fatto ricorso, e il presidente del TAR aveva sospeso l'efficacia di quel provvedimento di interdizione,

cosa succede? Che la partecipazione dei ministri Toninelli e Trenta, a questo punto, diventa irrilevante.

Rimane l'impossibilità di procedere allo sbarco senza l'indicazione del porto sicuro di sbarco. E che cos'è l'indicazione del porto sicuro di sbarco se non un atto (che non è atto politico)?

dagli adempimenti occorrenti per effettuare lo sbarco nel più breve tempo possibile, comportando il minore discostamento possibile dalla rotta e il minor aggravio per gli armatori. Quindi, la norma internazionale che è stata introdotta nell'ordinamento italiano, attraverso la ratifica della convenzione SAR, siglata ad Amburgo nel 1979, impone allo Stato italiano di indicare indicare il posto dove effettuare lo sbarco senza ritardo. Che cosa significa questo? Che non si tratta di un atto assistito dalla discrezionalità politica né di un atto assistito da ampia discrezionalità amministrativa; si tratta di un atto di discrezionalità tecnica, nell'ambito del quale, fermo restando che il se (l'*an*) non è in discussione, si può soltanto variare

la vicinanza del porto, l'organizzazione a terra quanto ad accoglienza e ordine pubblico. Questi sono gli elementi che possono variare l'indicazione (non concessione) del POS

pertenesse al Ministro dell'interno, in collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa. Il 12 febbraio del 2019 - scusate, ma non è stato detto - era stata attuata una modifica una modifica delle procedure operative *standard*. Tale modifica accentrava non più nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, come per i precedenti casi Diciotti e Gregoretti, la responsabilità dell'indicazione del POS, come correttamente afferma il tribunale di Palermo, poiché essa insiste immediatamente e - lo sottolineo - esclusivamente sul Ministro dell'interno. Quindi, tutto afferiva al Ministro dell'interno, tanto che il tribunale di Palermo esclude qualunque ipotesi di responsabilità anche del Capo di gabinetto del Ministro dell'interno, il prefetto Piantedosi.

dal punto di vista politico e scrive una lettera al ministro Salvini, invitandolo quantomeno a far venir meno

vi sono, in questa circostanza, elementi che qualificano la condotta e il comportamento del ministro Salvini come obiettivamente intesi a perseguire un preminente interesse pubblico qualificato

Ma che vuol dire? Con questa relazione, purtroppo, il presidente Gasparri fa ripiombare l'Italia all'epoca della Magna Charta Libertatum del 1215. Non è possibile, in uno Stato di diritto, affermare che se il Ministro

In quest'Assemblea non si devono verificare degli accordi di casta, come sembra evocato da qualcuno. Non bisogna accordarsi perché qui dentro, prima o poi, tocca a tutti.

voglio partire da una considerazione più volte ripetuta in quest'Assemblea, cioè che il Senato non è il giudice del ministro Salvini

però non posso non rilevare come in quest'Assemblea sia ritornato un argomento diventato di scottante attualità, ossia il rapporto tra la politica e la magistratura. Dal 1993, quando il Parlamento, sotto la spinta emotiva dell'opinione pubblica, ha eliminato la immunità parlamentare, non c'è il contrappeso al potere giudiziario e assistiamo frequentemente, reiteratamente, all'invasione di campo da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della politica, al di là del fatto che due *referendum* hanno stabilito la necessità di individuare la responsabilità civile dei magistrati e non se n'è mai più parlato.

considerazioni non possono allora non rilevare in questa discussione, che è l'unica forma non di corporativismo, ma di autotutela e di difesa delle istituzioni dall'invasione inopportuna della magistratura nei confronti della politica e dell'iniziativa politica. Questo è un argomento di cui dobbiamo tener conto e non soltanto come fa il presidente Renzi, che non perde occasione per citare la questione delle fondazioni, che evidentemente gli stanno particolarmente a cuore. Il problema è molto più generale e riguarda tutti; non può riguardare una parte o un singolo soggetto. I fatti sono stati enunciati in maniera puntuale dal relatore e sono stati ripresi. Il comportamento del ministro Salvini è stato quello di ottemperare ad un indirizzo politico che era stato stabilito (e non poteva essere diversamente ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione) dal Presidente del Consiglio nell'esercizio di questa sua espressione ha garantito il rispetto dei diritti umani, ha osservato le leggi, non ha abbandonato su un barcone degli immigrati, peraltro clandestini che non avevano titolo legittimo per entrare nel nostro Paese. Questa è la verità. Ha consentito l'evacuazione per motivi medici; ha consentito, nonostante non lo condividesse, lo sbarco dei minori non accompagnati, così come ha invitato a fare il Presidente del Consiglio, che fino a quel momento col suo silenzio aveva ratificato il comportamento del suo Ministro dell'interno. Considero quindi corretta la conclusione alla quale è arrivata la Giunta parlamentari, che ha individuato la sussistenza della seconda scriminante prevista dall'articolo 9 della legge cioè l'aver agito nell'esercizio della funzione di Governo e nel preminente interesse pubblico. Dobbiamo quindi verificare se nella fattispecie l'azione rientrasse nell'esercizio della funzione di Governo. Come ho detto prima, l'attività di coordinamento, di controllo del Governo è esercitata dal Presidente del Consiglio ed è stato ricordato che il 1° agosto 2019 il Ministro dell'interno ha agito di concerto col Ministro della difesa e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, quindi con un atto collegiale che è stato assentito dal Presidente del Consiglio.

i Ministri devono tenere in determinate circostanze; ci sono rapporti e contatti informali, ci sono consuetudini, ci sono assensi. Pertanto, l'aver agito in primo luogo in concerto con gli altri Ministri e l'aver portato avanti quella iniziativa con l'assenso, col silenzio assenso del Presidente del Consiglio qualifica assolutamente la funzione del ministro Salvini in quel momento come funzione di Governo, tanto è vero che quando il Presidente del Consiglio ha ritenuto di non condividere più un certo comportamento, per sue motivazioni che il ministro Salvini non ha accettato ma che ha rispettato (non poteva fare diversamente, visto che l'obbligo

far scendere i minori non accompagnati. Vi è quindi sicuramente l'esercizio della funzione di Governo, così come individuata e stabilita dal Presidente del Consiglio. Ora bisogna vedere se c'è il preminente interesse pubblico. Gli oratori che mi hanno preceduto dicono che non esiste. Che cos'è il preminente interesse pubblico? È la tutela e la salvaguardia di diritti non negoziabili dei cittadini del nostro Paese. Paese. In quelle circostanze di tempo e di luogo, l'Italia era diventata il porto naturale di attracco di barconi di extracomunitari, lo stiamo vivendo anche in questi giorni, non credo che la situazione sia mutata. Quell'atteggiamento è servito a convincere, al di là dell'accordo firmato nel 2018 sulla redistribuzione degli immigrati, che poi non è stato rispettato, tant'è vero che Malta, che era il Paese competente ad intervenire per la Convenzione internazionale, non lo ha fatto se non

nazionale, quello di garantire la giusta redistribuzione degli extracomunitari sul territorio europeo? 650.00 gli extracomunitari clandestini illegali che vengono mantenuti dal nostro Paese ancora oggi e che costano svariati miliardi di euro. In un momento di difficoltà che non è soltanto determinato dal Covid, ma che esiste da tempo, con cinque milioni di poveri non è un interesse preminente nazionale garantire la tutela dei diritti dei concittadini prima di aprirsi alla solidarietà?

e non mi meraviglio del fatto che il presidente Renzi non abbia cambiato idea rispetto alle altre richieste di autorizzazione a procedere. Mi meraviglio e mi fa decisamente specie, invece, che abbiano cambiato idea i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che addirittura in maniera appassionata avevano rigettato la richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti e che invece oggi hanno cambiato idea e probabilmente lo hanno fatto non su questioni in punto di diritto, ma soltanto perché ieri erano al Governo con la Lega e oggi invece la Lega è all'opposizione. Non è questo il modo di condurre le battaglie politiche. È questa, cari colleghi, l'unica sede nella quale possiamo gridare la nostra indipendenza nelle scelte politiche, la nostra prerogativa di fare determinate scelte politiche, di fronte alle continue invasioni di campo da parte della magistratura. I fatti recenti sono la prova di quanto da tempo qualcuno di noi va dicendo e che oggi trova altri proseliti. È un fatto oggettivo. Che si facciano le scuse *a posteriori*, a funerali celebrati, onestamente forse può servire a darvi un'attenuante alla coscienza, ma non serve sicuramente a ripristinare la verità e il rispetto dei fatti e delle istituzioni. Credo, colleghi, che non che non sia con le autorizzazioni a procedere che si conducono le battaglie politiche. Le battaglie politiche si conducono in quest'Aula, si conducono con il confronto delle idee, con il contributo dei cittadini e del voto e non certamente mandando a processo in maniera ingiusta e non opportuna un rappresentante prima del Parlamento e poi del Governo qual è stato il ministro Salvini. La cosa ancora più grave è che c'è fondato motivo di ritenere che non soltanto l'autorizzazione a procedere che viene richiesta, se concessa, sarebbe inopportuna e non coperta dalle garanzie costituzionali, costituzionali, ma che voi con questo atto, se lo accettate, mandate un cittadino italiano, un rappresentante della Repubblica, un ex Ministro davanti a un plotone di esecuzione. Questa è una vostra responsabilità, della quale darete conto alle vostre coscienze e ai vostri elettori.

che si inserisce, tra l'altro, in un complicato rimpallo di responsabilità e di competenze fra le varie autorità straniere che sono chiamate a rispondere. Il tutto in una cornice normativa nazionale e internazionale di difficilissima lettura

Di questo se ne è parlato, se ne è trattato, come hanno detto anche i colleghi e i fatti sono stati ampiamente riassunti nella relazione proposta dal presidente Gasparri.

non vi sono elementi idonei a sostenere in giudizio l'assunto per cui l'obiettivo primario della condotta di rifiuto del POS da parte del Ministro fosse proprio quello di privare i migranti della loro libertà di locomozione e pregiudicare il loro diritto alla salute e gli altri dritti fondamentali. Sta dicendo, cioè che non vi era l'intento, non

ministri conferma che esiste l'esimente di cui all'articolo 9, cioè il famoso, trito e ritrito (perché ormai penso che anche i nostri cittadini sappiano esattamente che cosa sia) perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio delle funzioni di governo. Il tribunale, infatti, dice che la condotta del Ministro è apparsa animata dalla finalità di contrastare gli ingressi irregolari nel territorio italiano e di contrapporsi attivamente alla mancata assunzione di responsabilità degli eventi migratori da parte di altri Stati dell'Unione europea. Lo sta confermando. Questa è una contraddizione nella quale pare proprio emergere che, a volte, va bene sostenere una tesi quando è contro Salvini, mentre va male nel momento in cui la devi sostenere a favore dello stesso Riteniamo di condividere tutto ciò che è stato illustrato dal relatore. È pienamente provato che vi sia questo perseguimento di preminente interesse pubblico. Perseguimento non significa tutela effettiva, significa che hai operato nell'intento di e in funzione di

Non occorre perché sembra di continuare a ripeterlo, ma possiamo richiamare benissimo quanto già sostenuto sia nel caso Gregoretti, sia nel caso Diciotti. È chiaro: c'era un coinvolgimento politico governativo del Presidente del Consiglio e di tutto il Consiglio dei ministri sulle decisioni riguardanti la politica migratoria. Non occorre ricordare tutti gli interventi del presidente Conte, che sono stati fatti qui in Senato, in sede di dichiarazioni programmatiche o nelle comunicazioni in vista dei Consigli europei. Ricordiamo anche gli interventi degli altri Ministri:

I Ministeri si sono costituiti davanti al TAR, per difendere il decreto del 1° agosto. Vi è poi un carteggio particolare fra il ministro Salvini e il presidente Conte, nel quale, chiaramente, il Ministro ha lavorato da Ministro e il Presidente del Consiglio ha lavorato da Presidente del Consiglio, ovvero si è applicato pienamente l'articolo 95 della Costituzione, per cui il Presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, mantiene l'unità di indirizzo, promuove e coordina l'attività dei Ministri. È stato disposto e richiesto lo sbarco di minori, con ciò, argomentando *a contrario*, ordinando o dando una direttiva sullo sbarco di altri.

Vi sono dei princìpi ai quali dobbiamo richiamarci, come ha detto anche il senatore Renzi, anche se si afferma la separazione dei poteri, poi però, nel momento in cui bisogna agire nei confronti Salvini, va bene agire nei confronti Salvini. Dobbiamo ricordare che vi è un'autonomia della politica e un'indipendenza della magistratura, ma, in conclusione, la vera questione è che l'avversario lo si combatte con i voti e non certo in un'aula di tribunale.

la discussione è proprio sulla possibilità di declinare delle politiche dure, radicali, forti sul fronte dei flussi migratori. Lo dimostra anche la distribuzione dei tempi, data dal Gruppo Misto. Chi difende la linea morbida, la linea del Governo, ha dieci minuti, chi invece, come me, prova a dire qualcosa di diverso, ne ha soltanto cinque;

si deve vedere un po' di cicatrice addosso ed è esattamente quello che si deve vedere rispetto alla vicenda di Salvini, che è uno degli interpreti della linea dura e quindi mandando a processo Salvini la seconda volta, si dice «voi non potete e non dovete avere nei Governi quella linea che con il primo Governo, con una maggioranza diversa, Salvini interpretò come Ministro dell'interno». Quello era comunque il Ministro dell'interno di un Governo cui io diedi la fiducia. Infatti fu salvato nel caso della nave Diciotti, anche dal MoVimento 5 Stelle che allora ovviamente aveva piattaforma Rousseau, aveva dato magari qualche Maalox a qualcuno che aveva mal di pancia, però alla fine fu salvato perché c'era la maggioranza da mandare avanti. È così o non è così? Certo che è così, poi cambiano le alleanze ed ecco che tutto diventa barattabile. È un po' come il MES; alla fine, tanto si è fatto, che l'hanno messo nero su bianco e doveva esserci perché va dato un segnale politico. Visto che la questione è squisitamente politica e cioè se è possibile avere una politica dura, ferma e decisa sul controllo dei flussi migratori, Bruxelles ci sta dicendo di stare attenti alle alleanze che facciamo perché altrimenti finisce che vi mandiamo a processo. terra, terra - la partita di cui stiamo discutendo. Non ci deve essere la possibilità che i Paesi abbiano una linea ferma sul controllo dei flussi migratori *(Applausi)* di qua, ci sarà chi dice basta con i flussi incontrollati delle migrazioni e, dall'altra parte, c'è chi chiude un occhio, c'è chi afferma di essersi accorto adesso dell'emergenza che arriva dalla Tunisia.

Esercito e Forze dell'ordine per andare a prendere quelli che facevano *running* sulla spiaggia. C'era uno isolato che prendeva il sole e si è ritrovato metà delle Forze dell'ordine per andarlo a prendere. Allora fateci capire un po', tutta questa roba che avete riuscite a controllare quelli che fanno *jogging* sulla spiaggia durante il *lockdown*, e non riuscite, con l'impiego satellitare, a tenere sotto controllo una parte di Mediterraneo? La gente ha capito che non vogliono farlo. Certo che non vogliono farlo, perché semplicemente l'Europa agisce su una doppia gabbia per disarticolare gli Stati e creare delle tensioni sociali; dall'alto, c'è la morsa che arriva attraverso il capitale finanziario e, dal basso, attraverso le migrazioni di massa. Così chiudi chiudi i Paesi, disarticoli gli Stati e crei delle tensioni che, guarda caso, si scaricheranno sempre, ancora una volta, sulle parti più deboli delle città e del Paese, sulle periferie già abitate da disoccupati, da gente invisibile rispetto alle politiche del lavoro, gente che - guarda caso - è costretta a vivere in condizioni di assoluto disagio

quindi dicendo che queste tensioni si scaricano sulle periferie che - guarda caso - sono i luoghi dove è più plastico e più evidente

costo. Finora nessuno ci ha creduto, a cominciare dalla sinistra che guarda caso ha perso i voti proprio in periferia perché è proprio lì il disagio di un'integrazione mai consumata,

si scarica, aumentando le tensioni sociali. È nelle periferie che ci sono le urgenze abitative. È nelle periferie che c'è un problema perché mancano i servizi, sociali, È lì il problema di fondo. Questo è il tema: vogliono accogliere e poi pensano che l'integrazione arrivi da sé. Stiamo vivendo un momento particolarmente

molto controllati, attraverso il *lockdown* e la privazione della libertà di circolare; dall'altra parte si assiste invece a degli strani ingressi incontrollati, a dei voli non controllati, a persone che rischiano di portare un possibile contagio.

perché Salvini, quando occupava il posto di Ministro, non lo occupava come un re, ma lo stava occupando da Ministro dell'interno di una delle due forze che componevano la maggioranza di quel Governo.

ed è questo il motivo per cui i pacchetti sicurezza alla fine hanno trovato una maggioranza; poi qualcuno tirava un po' da una parte e qualcun altro ha cercato di moderare, per l'amor del Cielo. Però quella maggioranza è stata trovata: quella voleva essere una linea comune. Adesso, cambiando il paradigma politico, quei decreti sicurezza imbarazzano e quello che ha fatto il primo Governo della legislatura imbarazza, però le tracce ci sono. Sui flussi migratori io penso che, con questo voto, si capirà in maniera plastica chi decide in un modo e chi decide in un altro. Con questo voto noi capiremo chi dice no a flussi migratori incontrollati, chi dice che qualcuno ci sta guadagnando e ci sta lucrando con certi flussi migratori e, dall'altra parte, chi invece

emergendo nella loro tensione, perché - come dicevo prima - quando non si riesce a controllare questi sbarchi, non si scaricano dei cittadini stranieri, ma si scaricano delle tensioni su altri cittadini. una volta e per sempre si prenda una linea. Credo che questa linea sia profondamente dettata dall'Europa: l'Europa, attraverso i flussi incontrollati e attraverso queste migrazioni di massa, vuole creare il panico all'interno dei Paesi europei. È un disegno preciso È un disegno preciso che hanno in Europa e questo disegno va smantellato. Ecco perché più di una volta ho suggerito di rompere la gabbia dell'Unione europea, perché dentro ci sono anche le tossine di quella che secondo me è una cattiva politica anche sui temi migratori: dall'alto con la finanza e dal basso con i

Signor Presidente, il 9 marzo 1977 Aldo Moro alla Camera, in un memorabile intervento sulla vicenda Lockheed, in difesa di Luigi Gui pronunciava queste parole: «C'è il rischio obiettivo di un'inammissibile politicizzazione e quello, altrettanto grave, che il nostro comportamento sia considerato inficiato da ragioni di parte, in una qualsiasi direzione». rischio che si corre ogni volta che una Camera è chiamata a decidere sull'autorizzazione a procedere di un suo componente. Per questo mi voglio attenere ai fatti, alle norme e alla giurisprudenza. Nella relazione del presidente Gasparri si afferma: «in questa sede non occorre valutare se siano o meno condivisibili le scelte effettuate dal ministro Salvini» ... «ma solo se queste ultime fossero rivolte o meno al perseguimento di un interesse pubblico inerente all'azione di Governo». La legge costituzionale n. 1 del 1989, recante norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione, definisce i due elementi essenziali il primo è l'esercizio di una funzione di Governo e il secondo è il perseguimento di un preminente interesse pubblico. Questi sono i parametri per valutare l'azione di un Ministro o del Presidente del Consiglio, che sono stati confermati da giurisprudenza costante della Cassazione (per citarne una per tutte, ricordo la sentenza n. 8854 del 1998). Il senatore Salvini ha perseguito un interesse pubblico preminente? Quale sarebbe? Nel caso della Open Arms l'interesse preminente era il dovere di soccorso e l'attracco a un porto sicuro. Sulla Open Arms ne sono state dette di tutti i colori - «è una nave spagnola», «è una nave privata» - ma il dovere di soccorso in mare opera per tutti.

Richiamando diverse convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia - che, voglio ricordare, sono fonti sovraordinate rispetto al diritto statale - la Corte ha dato una definizione molto estesa del dovere di soccorso in mare stabilendo che questo è inderogabile e può dirsi adempiuto solo con lo sbarco dei migranti, che deve avvenire nel più breve tempo ragionevolmente possibile in un luogo dove possono chiedere protezione internazionale, ovvero un'operazione che, secondo la Cassazione, non può certo essere effettuata sulla nave. A sostegno viene chiamata la risoluzione del Consiglio d'Europa 1821 del 2011, che stabilisce che luogo sicuro è quello dove viene garantita la protezione fisica delle persone, ma anche il rispetto dei loro diritti fondamentali. L'arresto di Carola Rackete è stato dichiarato illegittimo perché solo attraccando in banchina, anche contro il divieto di ingresso italiano, ha adempiuto fino in fondo al dovere di soccorso imposto dalla normativa sovranazionale applicabile. Si tratta di una pronuncia che mette al centro il dovere del soccorso del migrante, di fatto riducendo molto la linea che distingue i rifugiati dai migranti economici, per i quali la protezione internazionale non opera, stabilendo che prima di tutto bisogna consentire loro lo sbarco, dato che la valutazione dello *status* richiede tempo e non può essere certo fatta in mare. Il *focus* è la qualificazione giuridica della decisione di non autorizzare lo sbarco fino a quando non si è ricevuta la manifestazione di disponibilità da altri Stati europei alla distribuzione dei migranti. Bisogna dimostrare che, anche se è un atto rientrante nella funzione di Governo, il ritardo dell'autorizzazione allo sbarco deve essere originato da una situazione di pericolo per la sicurezza dello Stato e dei suoi confini e che questa situazione di pericolo sia stata prevalente nel bilanciamento dei diritti in conflitto, sul dovere di soccorso dei migranti e sulla tutela della loro dignità e libertà personale. La Costituzione, agli articoli 2 e 10, difende i diritti fondamentali e irrinunciabili. Le convenienze politiche del momento non possono sottomettere la cultura giuridica e la tutela della Costituzione a interessi di parte ed è di questo che stiamo parlando adesso. La giurisprudenza della Cassazione severa nello stabilire i confini del sequestro di persona: basta che la vittima, per un periodo anche breve, versi in condizione di impossibilità relativa e non assoluta di autoliberazione,

Il professor Filippo Sgubbi, che ha scritto cose fondamentali per il diritto penale, sostiene che il reato e la colpa sono uno stato che precede la commissione di un fatto. Non si tratta di una colpa generale inerente alla persona umana come tale, ma è legata al ruolo sociale ricoperto e alla tipologia di attività che svolge nella vita. Si badi bene, quindi: non a uno specifico fatto; ruolo e attività svolta. per cui sono stati trattenuti in mare per diciannove giorni. Ma lo pensava veramente oppure si trattava di una scelta tutta politica per perseguire fini politici di parte? La definizione più corretta è quella di uso populista della questione criminale, per garantire al potere che la esercita di acquisire il consenso popolare e placarne così la pressione o forse, meglio, per eccitarne la compulsione. Il popolo non è protagonista di una politica che accresce il suo ruolo, ma viene usato come destinatario di un messaggio legislativo o di Governo, il cui fine è quello di arginarne la pressione placandone le inquietudini con operazioni di pura facciata. Peccato che questa volta l'operazione non fosse di facciata, ma abbia assunto i contorni e la sostanza del sequestro di persona. Orazio in un suo *carmen*, le parole «*integer vitae scelerisque purus*», scrive che chi è integro di vita e puro di colpa non ha bisogno di strali, né dell'arco, né della faretra colma di frecce avvelenate. Sembra scritta per il senatore Salvini, gran maestro nel seminare veleni politici. Ma in uno Stato di diritto, quale noi siamo, c'è sempre un momento in cui il diritto prevale sui veleni e sulla propaganda. diceva infatti Aldo Moro: «al di là del cinismo opportunistico», «una legge morale, tutta intera, senza compromessi, abbia infine a valere e dominare la politica». Una legge morale per la politica. Questi sono i motivi forti che stanno sotto il voto che siamo chiamati a dare oggi, ed è per questo che io voterò a favore dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini.

Signor Presidente, come ricordavano molti colleghi prima di me, è la terza volta che ci occupiamo sostanzialmente della stessa questione (Diciotti, Gregoretti e oggi Open Arms), ma alla fine, pur con alcune particolarità e specificità, il tema è sempre quello. La maggioranza dice che non spetta al Senato ergersi a giudice e stabilire se c'è stato o non c'è stato un reato nel comportamento del ministro Salvini. La collega Bonino dice non siamo noi che dobbiamo trasformarci in uno scudo dal processo per il senatore Salvini. Ebbene, cari colleghi, non è proprio così, perché noi in questo momento svolgiamo anche una funzione giurisdizionale. È vero che non spetta a noi giudicare se è stato commesso o no un reato, ma spetta certamente al Senato stabilire se esiste o non esiste l'esimente speciale di cui alla legge costituzionale. E su questa esimente speciale possiamo giudicare soltanto noi. La magistratura ordinaria non può entrare nel merito di questa specifica questione sulla quale, ripeto, il Senato deve pronunciarsi esercitando una funzione giurisdizionale. Noi in questo momento siamo giudici *(Applausi)*; anche se parliamo di politica, siamo giudici e dobbiamo stabilire se esiste o non esiste il perseguimento di un preminente interesse pubblico nella funzione di Governo esercitata dal ministro Salvini quando prendeva le sue decisioni. I colleghi della maggioranza dicono il preminente interesse pubblico non c'era e posso capirli: chi nega il valore dell'identità nazionale, nazionale, e della sicurezza e dei confini, chi vorrebbe un mondo senza confini, in cui siamo tutti consumatori, senza identità, senza cultura e senza specificità, posso capire che non comprenda il valore di un preminente interesse nazionale nel difendere i confini da un'invasione

ci vogliamo prendere in giro, cari colleghi della maggioranza? Ma quali profughi? L'altro giorno uno è sbarcato addirittura con il barboncino, come dire: «Mi piace l'Italia, ci ritorno, anche se ho il decreto di espulsione, tanto ho l'albergo gratis e tutto quello che mi serve; mi rimpatriano prima o poi gratis e poi ritorno». Forse al massimo di coloro che arrivano sulle nostre coste sono davvero profughi: tutti gli altri sono migranti economici, nella migliore delle ipotesi, perché, dentro quella massa di disperati, ci sono anche i delinquenti, gli esponenti della mafia nigeriana e ci sono anche le vittime, di cui voi anime belle della sinistra, quando si discute di questi argomenti, vi scordate sempre ci sono le ragazze destinate alla prostituzione, ci sono giovani destinati allo spaccio e ragazzotti ben nerboruti destinati a gestire le piazze dello spaccio per conto delle mafie africane e via di questo passo, ma di tutto questo non si deve e non si può parlare. però, non è qui il preminente interesse pubblico, io direi l'assoluto interesse nazionale, dov'è? Ma come si fa a negare che la massa di disperati che arriva in Italia e che noi accogliamo a braccia aperte, alla fine, nella migliore delle ipotesi, diventa oggetto oggetto di sfruttamento del lavoro nero, quindi concorrenza sleale nei confronti dei lavoratori e degli imprenditori onesti? Come si fa a negare che diventa manovalanza per la delinquenza, che diventa oggetto di sfruttamento della prostituzione va a riempire le nostre carceri va a competere con gli italiani che hanno diritto alla minima assistenza (che gli viene sottratta da chi invece non ne ha diritto perché non essendo profugo non ha diritto di stare sul suolo nazionale)? Come si fa a negare che qui vi sia un interesse nazionale e non solo un interesse pubblico? Eppure, per ideologia voi lo negate, perché non avete perso l'antico vizio di abbattere l'avversario per via giudiziaria, quando non riuscite ad abbatterlo per via politica. Questo è il vero dibattito che oggi stiamo facendo, che non c'entra nulla con la funzione giurisdizionale che invece dovremmo svolgere.

da noi si può permettere di dire quello che vuole. Dice il senatore Renzi che non si blocca l'immigrazione tenendo un barcone in mezzo al mare. caro senatore Renzi, guardi che i dati la smentiscono. Quando il ministro Salvini, con i suoi limiti, cercava di tenere lontana l'ondata di invasione dalle nostre coste, in un anno sbarcavano 3.000-3.500 migranti: oggi siamo a quattro volte di più. C'è da dire che è stato lungimirante il ministro Salvini diceva il ministro Salvini, ma lo diceva il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, già il 13 giugno

Soprattutto oggi stiamo verificando un'altra questione, che veramente ci deve allarmare: in mezzo a questa nuova massa di migranti che sta arrivando, ci sono purtroppo tante persone positive al Covid-19, centinaia e centinaia

almeno 600 positivi finora accertati. li vuole ospitare nel suo Comune, penso che troverebbe qualche obiezione anche da parte dei suoi concittadini. Ebbene queste persone sbarcano e poi vengono lasciate scappare; vengono lasciate scappare e non si sa dove vanno. Non c'è un pericolo per la sanità pubblica in questo caso? Non c'è. Non c'è, perché per ideologia voi lo volete negare. Solo per questo non c'è. Ma il ministro Lamorgese (che se non sbaglio è Ministro dell'interno e qualche competenza e qualche potere potrebbe averli in questa materia) dice che la situazione degli sbarchi è inaccettabile. Lo dice il ministro dell'interno Lamorgese. Se è allora inaccettabile oggi, non lo era quando il ministro Salvini faceva quello che faceva per difendere i confini nazionali? Anzi, come ho detto più volte in quest'Aula e lo ripeto, caro senatore Salvini, lei una cosa in più avrebbe potuto farla, secondo noi,

e per evitare i morti in mare. Infatti, l'unico modo per evitare i morti in mare è impedire che partano, non bloccarli a metà strada o bloccare i porti italiani: impedire che si muovano dai porti dell'Africa. Questo bisognava veramente fare. Ma capisco che, con la maggioranza raffazzonata di allora, sarebbe stato impossibile ottenere una cosa del genere. Ma oggi il ministro Lamorgese dice che

è la terza volta in meno di due anni che il Senato è chiamato a valutare un'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini. Ci fu il caso Diciotti, poi quello della nave Gregoretti e ora l'Assemblea esamina gli eventi che coinvolsero la Open Arms nell'agosto dello scorso anno. I reati che gli sono stati contestati dalla procura della Repubblica sono il sequestro di persona plurimo, aggravato dall'essere stato commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, anche in danno di minori, nonché il delitto di rifiuto di atti d'ufficio. Ancora una volta - è bene ricordarlo - non dobbiamo discutere delle eventuali responsabilità penali dell'allora Ministro dell'interno, ma solamente se le sue azioni sono riconducibili a una delle esimenti previste dalla legge costituzionale n. Il Senato deve dunque decidere se Salvini agì per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per perseguire un preminente interesse pubblico. Abbiamo ascoltato la relazione del presidente Gasparri, sulla quale esprimemmo in Giunta un voto contrario, altri hanno già ricostruito nei dettagli la catena di eventi che si sono succeduti tra il 1° e il 20 agosto. Per questa ragione mi concentrerò soltanto su quegli elementi cruciali che, a mio giudizio, qualificano in maniera chiara le azioni dell'ex - per sua scelta - Ministro dell'interno, ai fini del giudizio cui il Senato è chiamato. In primo luogo, è opportuna una riflessione sul divieto di ingresso imposto alla Open Arms con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa e dei trasporti. Tale provvedimento, che si basa sul decreto sicurezza - *bis*, teorizzava un'ipotesi di passaggio non inoffensivo della Open Arms e faceva riferimento a un generico pericolo di natura terroristica per il nostro Paese. I legali della ONG spagnola presentarono un ricorso urgente al TAR, che venne accolto il 14 agosto e che sospese in via cautelare gli effetti del provvedimento interministeriale. In alcun modo risulta - così come sostenuto dall'allora ministro Salvini - che il TAR abbia accolto parzialmente il ricorso della Open Arms. Nella motivazione, invece, si rigetta l'ipotesi di passaggio non inoffensivo che era stata posta alla base del decreto interministeriale e si prospetta una situazione di eccezionale gravità e urgenza a bordo della Open Arms, che da sola giustificava l'ingresso della stessa nelle acque territoriali del Paese. Qualora sorgessero dubbi interpretativi, giova ricordare che, a seguito della sentenza del TAR, la proposta del Ministro dell'interno di disporre un secondo provvedimento non ricevette il supporto indispensabile degli altri Ministri. Da ciò si può facilmente dedurre come, non essendoci accordo tra i Ministri competenti, non si può certamente qualificare come atto di Governo la successiva attività del ministro Salvini che operava in relazione alle proprie attribuzioni di Ministro dell'interno. Dal momento in cui viene quindi sospeso il divieto di ingresso imposto alla Open Arms il 14 agosto e la nave fa il proprio ingresso nelle nostre acque territoriali, è inconfutabile che l'Italia abbia l'obbligo del rilascio del POS, dell'indicazione del posto sicuro dove attraccare. È un atto dovuto di cui è esclusivo responsabile il Ministro dell'interno. È bene ricordare che fu proprio il Ministro dell'interno che, nel tavolo tecnico di coordinamento del contrasto all'immigrazione illegale via mare, il 12 febbraio 2019 stabilì di togliere la competenza al capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e affidarla - guarda caso - al capo di gabinetto del Ministro, alle dirette dipendenze dello stesso Salvini. L'intenzione era chiara: usare l'indicazione del POS come strumento politico, cosa chiaramente in contrasto con la normativa internazionale, che invece lo qualifica come l'atto conclusivo dovuto di ogni operazione di salvataggio in mare. Anche per tale considerazione non è assolutamente condivisibile la posizione sostenuta da Salvini e da Gasparri, che ritengono invece la responsabilità collegiale del Governo per giustificare il preminente interesse pubblico. A tal proposito, è utile ripercorrere brevemente il carteggio intercorso in quei giorni tra il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'interno. Il 14 agosto, il presidente Conte, avendo ricevuto informazioni che confermavano la presenza a bordo di alcune decine di minori in condizioni di emergenza e in pericolo di vita, invitava il Ministro dell'interno ad adottare con urgenza i provvedimenti necessari per assicurare la loro assistenza e tutela, così come previsto dalle norme internazionali cui l'Italia si uniformava e si uniforma. Si badi bene, questa è un'attività indipendente dall'indicazione del POS per gli altri naufraghi. Il giorno seguente il ministro Salvini osservava sostanzialmente che si trattava di presunti minori non accompagnati e, inoltre, che, non essendo presenti sul territorio nazionale, poiché la nave non era al momento al momento della nota del 14 agosto in acque territoriali, la competenza a tutelarli spettava semmai alla Spagna, come Stato di bandiera della Open Arms. Il giorno seguente il presidente Conte inviava a Salvini un'altra nota in cui si discostava fortemente dalle considerazioni sulla presunzione di affidamento di minori ad altri migranti presenti sulla nave e in cui dimostrava la contrarietà alle tesi del ministro Salvini. Nella stessa nota il *Premier* sottolineava come fosse indifferibile l'incombente giuridico, oltre che umanitario, dell'autorizzazione allo sbarco immediato dei minori indipendentemente dalla redistribuzione verso altri Stati europei. Conte evidenziava come, comunque, Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna si erano già dimostrati disponibili a condividere l'ospitalità di tutte le persone a bordo. il presidente Conte sottolineava come si fossero anche verificate quelle nuove condizioni per il rilascio del POS concordate in occasione del tavolo tecnico sul contrasto all'immigrazione illegale e che hanno comportato modifiche alla direttiva SOP 009/15, nel senso che il POS potesse essere rilasciato solo dopo l'attivazione delle trattative per la distribuzione dei migranti tra i Paesi europei. In altre parole, visto che c'era la disponibilità dei Paesi europei non vi era più ragione di impedire lo sbarco. Solo il 17 agosto Salvini cedeva e faceva sbarcare "suo malgrado" i minori, manifestando chiaramente, per iscritto, al Presidente del Consiglio dei ministri di non condividere le motivazioni e le responsabilità dello sbarco. Nelle comunicazioni intercorse tra i due emerge con chiarezza come il Presidente del Consiglio dei ministri sia intervenuto senza alcuna sostituzione del Ministro e per riparare all'evidente inadempienza del suo Ministro dell'interno. Quindi, nessuna collegialità, ma l'azione solitaria del Ministro che ha trasformato un atto dovuto (come lo sbarco dei minori), previsto dalle convenzioni internazionali, anche questo - di contrasto all'immigrazione, per di più subordinato alla redistribuzione a livello europeo. Da ultimo, è opportuno riflettere sulla posizione del comandante della Open Arms. Come noto, il comandante di una nave ha precisi doveri e responsabilità, come previsto dall'articolo 295 del codice della navigazione, tra i quali riveste particolare importanza la tutela dell'ordine e della sicurezza a bordo. In quei giorni l'Open Arms arrivò a ospitare più di 160 persone a bordo, tra equipaggio e naufraghi, e in condizioni meteorologiche difficili.

mettendo a repentaglio la loro vita. È in questo difficile contesto che il comandante matura la convinzione di non poter garantire la sicurezza a bordo qualora i naufraghi salvati nel terzo evento SAR fossero stati sbarcati in via preferenziale a Malta. Difficile, infatti, immaginare che gli altri che stavano da più giorni in balia delle onde avrebbero compreso la differenza di trattamento, anche in considerazione della paura di essere rimpatriati nei centri di detenzione libici e magari fatti oggetto di armi da fuoco. Lo stesso vale per la proposta, rifiutata, di proseguire la navigazione fino alla Spagna. L'Open Arms non era affatto attrezzata per proseguire in sicurezza il viaggio e le persone a bordo erano ormai stremate. Come ha ben argomentato la terza sezione penale della Corte suprema di cassazione nella sentenza del 16 gennaio 2020, n.

accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro, nel cosiddetto *place of safety* (POS). Per tutte queste ragioni

Presidente, colleghi, il presidente Grasso ha esposto molto bene una serie di questioni e vorrei riprenderne alcune. ascoltando gli interventi nel corso della mattinata avrei cambiato l'ordine degli argomenti e, invece di parlare per primo della ragion di Stato, sulla quale soffermerò, partirei dal titolo di questa giornata e di queste nostre riflessioni, che è «Le persone sono strumenti o sono fini?» Le persone sono fini secondo la nostra Costituzione, ma prima ancora secondo la nostra umanità,

dalla fede, è una cultura della quale siamo permeati. Le persone sono quindi strumenti o sono fini? Ho sentito parlare di difesa dei confini e di quant'altro, ma se le persone non sono strumenti e sono fini mi chiedo di cosa stiamo parlando qui oggi. Continuiamo a confrontarci con la difesa dei confini quando il fatto con cui ci confrontiamo è che c'erano delle persone soccorse in mare, naufraghi richiedenti asilo e richiedenti soccorso che avevano diritto al completamento del soccorso. Decidiamo come incasellare questo punto e lo vediamo subito. Per comodità penso che sia giusto ricordare alcuni fatti inconfutabili e contestare alcune

(mentre era omologata per 19), con un equipaggio ormai esausto e con due bagni alla turca a bordo

accertate dai medici che salirono a bordo e poi successivamente verificate anche dal procuratore della Repubblica di Agrigento. Si trattava cioè di un

che cosa sono le persone e qual è il metro di giudizio delle sofferenze che si possono infliggere. E poi vedremo la ragion di Stato. C'è una misura? E da cosa dipende? dipende? Dalla cittadinanza? Dalle condizioni? O non è uguale per tutte le persone la misura della sofferenza? O forse c'è qualcuno che si può far soffrire un po' di più? più? Questo si sta dicendo. La situazione era esasperata al punto che alla sola idea di poter essere riportati in Libia - perché di questo stiamo parlando - alcuni si gettarono in mare non sapendo nuotare. Le condizioni metereologiche erano disastrose

che l'ammiraglio capo delle capitanerie di porto scrive al Capo di gabinetto dicendo che aveva autorizzato personalmente la vicinanza e l'ancoraggio a Lampedusa perché le condizioni meteorologiche erano proibitive e non avrebbe autorizzato altri porti perché c'era pericolo. Mi rivolgo soprattutto

anche sui nemici sconfitti: dopo che si è affondata la loro nave, li si va a soccorrere. E lo dico se vogliamo richiamarci a qualche nobile tradizione, perché l'Italia di nobili tradizioni ne ha moltissime.

cautelare che fa decadere il decreto con cui si proibivano l'ingresso e lo sbarco nel porto. L'autorità giudiziaria, proprio per l'indipendenza tra la politica e la magistratura, non può imporre e ordinare di sbarcare, perché quello è l'atto di alta amministrazione del Governo e del Ministro. Toglie efficacia al tuo provvedimento e poi sei tu che devi provvedere. A quel punto, il ministro Salvini ha provato a fare un altro decreto che - guarda caso - il Ministro della difesa si è rifiutato - a proposito di collaborazione del Governo - di sottoscrivere. D'altra parte, nell'idilliaca amorosi sensi sulle politiche di Governo di quell'agosto del 2019 non penso che possa sembrare strano. Anche la questione del cortesemente a mettere da parte e la difesa di Open Arms ne chiede una reiterazione per avere un'ulteriore specificazione e uno strumento, ma questo rientra nelle questioni difensive e a noi non interessa. Passiamo allora alla ragion di Stato.

e uno sforzo di arrampicamento sugli specchi che denotano una debolezza delle argomentazioni. Mentre nelle prime ipotesi sulla Diciotti si sosteneva che c'era stata una piena condivisione (nelle dichiarazioni pubbliche), qui si ricorre ad un interessante strumento giuridico istituzionale, e cioè che, se non c'è un atto esplicito che interviene autoritativamente sul Ministro - il quale aveva accentrato peraltro su di sé ogni provvedimento e potestà con i famosi decreti sicurezza

guardando al bene primario che è la libertà, hanno voluto disciplinare proprio il rapporto tra la legge che tutti devono osservare e quella potestà di scelta di scelta nell'interesse superiore nazionale, che solo eccezionalmente consente di violare e bypassare i limiti. Lo abbiamo visto

qui entrano in gioco le diverse concezioni del rapporto tra Stato e cittadino, la propaganda, il populismo e l'autoritarismo - si sarebbero violati i confini completando il soccorso? In che cosa sarebbero stati una minaccia? O forse si vuole velatamente e ipocritamente dire

forse affronta anche il rischio di affogare e i 40 gradi all'ombra. Siamo noi che non possiamo sopportare di fargli patire sofferenze del genere. La ragion di Stato che cos'è? La questione dell'immigrazione è puramente incidentale. Non basta affermare che vi è un generico fine politico e che con qualsiasi mezzo lo si può raggiungere perché allora,

responsabilità di mettere in campo, per quanto ci riguarda, sperando in un dialogo costruttivo anche con l'opposizione, un vero piano di gestione dei flussi migratori e del soccorso delle persone in cerca di asilo; un piano compiuto che veda anche l'Italia protagonista dello scenario internazionale. Prima gli italiani non vuol dire l'Italietta dei carrarmati di cartone che non conta niente né in Europa, né nel mondo, ma vuol dire conoscere la situazione internazionale, essere protagonista e misurarsi anche con gli ultimi avvenimenti che sono già diversi

molto privato. *(Commenti)*. Le voglio chiedere e voglio chiedere a tutti voi se ci siamo mai domandati quale sommessa preghiera vi fosse per quell'uomo che aveva il proiettile nel piede, per quelle donne che sono state violentate, per chi fuggiva dalle torture.

nell'anima? *(Proteste)*. Avete di fronte non gli scafisti, ma quelle persone! Per affrontare gli scafisti bisogna mettere in dubbio rapporti nazionali e internazionali e andare a discutere con Orban! è il coraggio che si chiede a chi vuole difendere gli italiani e a chi vuole legittimamente pregare per un mondo migliore.

Credo che avremmo potuto saltare molte valutazioni, se avessimo dato un'occhiata anche alle argomentazioni che sono state prodotte in sede di domanda di autorizzazione a procedere

stata fatta una sorta di operazione di ritaglio, per cercare di andare a definire puntualmente, con il cesello, ciò che può essere concepito come interesse pubblico e come funzione di Governo.

non posto in essere, e cioè l'omissione del ministro Salvini, secondo la richiesta di autorizzazione a procedere.

facendo però un po' di acrobazie: questo ha fatto il ministro dell'interno Salvini in quelle circostanze. L'interesse pubblico era volto a trovare una collaborazione fra gli Stati per la tutela e la salvaguardia di quelli che sono dei diritti inviolabili. Quindi, non c'è stata alcuna omissione; al contrario, sempre nell'autorizzazione a procedere, si legge chiaramente che il Ministro era impegnato nei tavoli proprio per individuare una soluzione.

che abbiamo controllato: quando si parla della questione relativa alla collegialità dell'atto

Detto questo, vorrei però soffermarmi adesso su alcune questioni che

collaborazione fra gli Stati nel momento in cui ci sono migranti da collocare, e l'atto di impugnazione sottoscritto dagli altri Ministri - sono esaustivi da un punto di vista giuridico. Prova ne è a tal proposito

della questione di ciò che ha fatto Salvini quando era Ministro dell'interno. Si tratta di una sorta di abbonamento, di tagliando, ma, in questo caso, il tagliando ha delle differenze rispetto a quelli precedenti. La differenza fondamentale - a mio avviso - è la questione che è scoppiata con riferimento alle famose *chat* di Palamara di cui nessuno vuole parlare. *(Applausi).* Noi siamo di fronte ad una situazione che

è che quanto è successo al nostro Presidente, testimoniato tra l'altro dagli ultimi fatti che sono emersi, non ha insegnato a nessuno quanto può essere grave la persecuzione giudiziaria; non lo ha insegnato a nessuno. *(Applausi)*. Io non sono qui per ascoltare qualcuno che dice

Ma questo non toglie che c'è una responsabilità politica sulle nostre spalle: il quadro che è emerso, di fronte al quale ancora non sono stati assunti provvedimenti da parte della politica

La questione dei migranti in questo Paese non è solo un interesse pubblico, ma è anche un allarme sociale che riguarda le persone. Nella mia piccola Regione li hanno portati di soppiatto, senza avvertire i sindaci, e li hanno fatti anche scappare;

l'occasione di oggi ci dà la possibilità di ricordarlo a noi tutti. *(Applausi)*.

Signor Presidente, innanzitutto rivolgo un pensiero alle nostre Forze dell'ordine, che, anche in questi minuti, stanno lottando per difendere i confini. Si sono infatti arruolati per difendere i confini non per fare da tassisti a ragazzotti con cappellini, telefonini e barboncini. Ringrazio la Guardia costiera per quello che fa. di riuscire ad avere dieci minuti di attenzione. Tanto si è già capito che il voto è politico. Proviamo tuttavia a entrare nel merito. Ringrazio il Governo per la sua abbondante presenza. *(Applausi)*. Non era dovuta, ma, se la forma è sostanza, ringrazio i banchi vuoti del Governo, che dimostrano il rispetto per quest'Aula. Noto l'abbondante presenza dei senatori a vita e mi riconfermo nell'idea che questa sia una figura ampiamente superata nelle nostre istituzioni. *(Applausi)*. Noto il fatto che non sia intervenuto nessuno del MoVimento 5 Stelle, e ciò evidentemente sottolinea l'imbarazzo. Ma devo dire che preferisco il bel tacer del MoVimento 5 Stelle alle gratuite supercazzole di Renzi e compagnia.

Entriamo nel merito. Sostengo l'iniziativa annunciata pochi minuti fa dal sindaco di Treviso, Mario Conte, che chiederà i danni al Governo italiano perché 129 immigrati presenti nella caserma di Treviso sono risultati positivi al Covid Treviso è il primo focolaio in Italia. Invece di prorogare stati di emergenza in carenza di emergenza, provvedete a evitare di far sbarcare gente che poi porta il contagio in giro per l'Italia. Se riparte il contagio, saremo noi a denunciare qualcuno che ha permesso che l'Italia corresse questo rischio. Inseguono gli italiani con le mascherine e poi fanno sbarcare centinaia di persone potenzialmente infette sulle spiagge danneggiando il nostro turismo. l'articolo 52 della Costituzione, la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Di tutta questa vicenda l'unica cosa di cui mi rammarico sarà il fatto di dover spiegare stasera e domani mattina ai miei due figli che papà andrà a processo non perché è un delinquente, ma perché ha fatto semplicemente il suo dovere da Ministro e da cittadino di questa Repubblica. Delle critiche politiche mi frega men che zero; di dover dare risposta ai miei due figli, invece, mi interessa un po' di più. E voi avete la responsabilità di questa spiegazione. So che per voi conterà poco, ma è l'unico peso che realmente mi porto dietro. Ho sentito tante cose prive di fondamento. Se dovessi riassumere

tratta di una nave pirata che il 1° agosto raccoglie degli immigrati in acque libiche e il 2 agosto raccoglie immigrati in acque maltesi. È una nave che ha diritto ad avere a bordo 19 immigrati e che arriverà ad averne più di 150. Se c'è qualcuno che ha commesso un crimine e ha messo a rischio la vita delle persone, è il comandante di quella nave pirata e non un Ministro che ha difeso il suo Paese. Il 1° agosto è in Libia 2 agosto a Malta. Poi entriamo su «Scherzi a parte». La nave chiede un porto sicuro a Malta e alla Spagna. Una nave spagnola acque maltesi non chiede un porto sicuro alla Finlandia, al Venezuela o all'Italia. Una nave spagnola chiede un porto sicuro alla Spagna e, siccome è in acque maltesi, a Malta. Malta e Spagna dicono: no, grazie; ci vediamo la prossima volta. Il 4 agosto Malta dice: da noi no. Il 9 agosto il comandante della nave pirata raccoglie altri 39 immigrati in acque maltesi, mettendo a rischio altre 39 persone. Malta dice: almeno questi 39 li faccio sbarcare a Malta. Lui, però, si rifiuta. Il 12 e il 14 agosto il comandante della nave scrive all'ambasciata spagnola a Malta. La nave spagnola scrive all'ambasciatore spagnolo a Malta. L'Italia non c'entra un fico secco. Sempre il 14 agosto,

inizia ad agitarsi, a fronte del mare mosso e di un comandante criminale a bordo di una nave pirata, diciamo di entrare nelle nostre acque territoriali fino a che la tempesta non passa, vietando con la capitaneria di porto, che dipendeva da un altro Ministro, espressamente l'ingresso nel porto. E contestualmente facciamo scendere migranti in condizioni mediche precarie. Il 17 agosto facciamo scendere ventisette presunti minorenni, nove dei quali poi si dimostreranno tutt'altro che minorenni. Quindi il "sequestro" è abbondantemente in corso e il Presidente del Consiglio evidentemente è assolutamente complice di questo eventuale reato, che non esiste. Il 18 agosto arriviamo veramente al surreale: dopo diciotto giorni la Spagna si sveglia e mette a disposizione un porto spagnolo. Il comandante della nave pirata ci pensa un po' e dice che è troppo lontano. Il 19 agosto la Spagna offre un porto più vicino, alle Baleari: bello, accogliente, località di villeggiatura. Il comandante ci pensa un po' e dice no no anche alle Baleari. Il 20 agosto, in pieno "sequestro", la Spagna manda una nave per accogliere gli immigrati in Italia e portarli in Spagna: no anche a questo. Il 19 agosto, in pieno sequestro teorico in corso, l'ex ministro Toninelli, attualmente senatore, rilascia un'intervista a «la Repubblica»: «I migranti li portiamo in Spagna con la Guardia costiera». No anche a questo. Era evidente il fatto che si trattava non di un naufragio, ma di una voluta invasione di campo e di una voluta violazione della legge. Ma lo capisce anche un bambino di sei anni. Dico questo con la massima tranquillità: se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee e a difendere le sue idee fino in fondo, o non valgono niente le sue idee o non vale niente lui. E io andrò fino in fondo, senza chiedere aiutini a nessuno. I numeri di Frontex dicono che, dopo il nostro pericoloso Governo, l'unico Paese in cui si sono moltiplicati gli sbarchi quest'anno è l'Italia: sbarchi dimezzati in Grecia, sbarchi dimezzati a Malta, sbarchi dimezzati in Spagna, sbarchi triplicati in Italia. Quindi, qualcuno dovrà pagare e non dico giudiziariamente, perché la differenza di cultura tra un liberaldemocratico e qualcuno che guarda a sinistra è che noi alle idee contrapponiamo altre idee *(Applausi)*, e non i tribunali o i processi politici. Ripeto: alle idee contrapponiamo altre idee. ho combattuto e combatterò le politiche sbagliate di Monti, della Fornero, di Renzi e della Azzolina, ma non li porterò mai davanti a un tribunale. L'unico tribunale è quello del popolo *(Applausi)*, del voto dei cittadini, degli elettori. In democrazia dovrebbe funzionare così. Mi avvio alla conclusione. Faccio presente che, fra i poveri naufraghi sbarcati quest'anno, le due nazionalità preponderanti sono quella tunisina, con più di 5.000 arrivi, e quella bengalese, con 2.000 arrivi.

economica che, in un momento di crisi che entra in milioni di case di cittadini italiani, mi convince ancor più che prima sia un dovere aiutare i cittadini italiani e poi occuparsi del resto del mondo. *(Applausi)*. Prima ho non il diritto, ma il dovere di trovare una casa, un lavoro e un posto in ospedale ai miei concittadini, che mi pagano lo stipendio. Potrei andare avanti a lungo. In ogni caso, torno a casa a testa alta, con un processo, ma a testa alta. perché alcuni di voi me lo dicono nei corridoi, me lo dicono alla *buvette*, me lo scrivono col messaggino: «Matteo, hai ragione, ma l'indicazione del partito è A me i messaggini o le chiacchiere da corridoio interessano men che zero. A me la giustizia alla Palamara interessa men che zero. *(Applausi)*. Io guardo i fatti. Io vado tranquillo in quei tribunali: ho già il primo appuntamento il 3 ottobre a Catania, mentre l'altro sarà a Palermo e sarà per me una gioia andare nella splendida terra di Sicilia per rimarcare il mio diritto e dovere a difendere la bellezza della nostra terra. Sono sicuro che la stragrande parte della magistratura sia composta da persone sane,

Ricordando che, non un sovranista, ma Einaudi diceva che, quando la politica entra nella giustizia, la giustizia esce dalla finestra, questo Paese, senza una profonda e sana riforma della giustizia, con una separazione delle carriere, con processi in tempi brevi e con la responsabilità per chi sbaglia sulla pelle dei cittadini, non sarà mai libero, moderno ed europeo. Vi ringrazio per la vostra scelta, che va al di là della realtà, delle date, dei fatti e delle evidenze, perché mi dà ancora più forza, più energia e più voglia di ribadire il diritto-dovere di amare il nostro Paese. Se qualcuno pensa o pensava - ho sentito anche gli interventi di questa mattina - di mettere paura a me,

E ogni riferimento al processo politico contro la Lombardia e i lombardi, ignorando quello che è accaduto a Roma e nel Lazio, è puramente voluto. Da una parte, si indaga su una donazione e, dall'altra, si fa finta di niente su 14 milioni di euro pubblici pagati per mascherine mai arrivate, ma il tempo è galantuomo. Io vi posso dire, e concludo ben sapendo quale sarà il verdetto di quest'Aula, che ci ritroveremo fra sei mesi, un anno, dieci anni. Oggi si manda a processo Salvini, un processo politico: mi sembra assolutamente evidente. Domani - ve lo dico la ruota gira, quando toccherà a qualcuno di voi - perché toccherà a qualcuno di voi - la Lega starà dalla parte delle garanzie e della libertà del Parlamento e dei cittadini. Non vi manderemo in un'aula di tribunale: saranno i cittadini a giudicarvi, e non i giudici. Capiterà a qualcuno di voi e la Lega starà dalla parte della libertà e delle garanzie, e non con le chiacchiere, ma con i fatti, col voto, a testa alta, con la schiena dritta. *(Applausi)*. Ringraziandovi Ringraziandovi quindi per quello che è evidentemente un processo politico, ringrazio anche i milioni di italiani - la maggioranza silenziosa, operosa e laboriosa - che chiedono un'immigrazione utile, limitata, positiva, controllata e qualificata. Il mio orgoglio da Ministro, sequestratore per qualcuno, è che, grazie al controllo dell'immigrazione clandestina, abbiamo più che dimezzato i morti nel mar Mediterraneo. *(Applausi)*. I tifosi dei porti aperti hanno le mani sporche di sangue e hanno trasformato il Mediterraneo in una fossa comune. Quindi io vi posso dire, con serenità, gioia e tranquillità, ricordando un grande italiano a cui non sarei degno neanche di allacciare le scarpe, che «chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola». Sono orgoglioso di rappresentare, con tutti i miei e i nostri difetti, l'Italia che ha portato arte, bellezza e cultura nel mondo, che non ha paura e vuole che vengano difesi la sua storia, i suoi confini, il suo onore e la sua dignità. Viva l'Italia. Viva la libertà. Viva la democrazia! Grazie a tutti coloro che mi manderanno a processo, perché mi fanno un gran regalo. In quel tribunale, a differenza di tanti, ci vado a testa alta e con la schiena dritta.

riprenda con le telecamere: non si può fare, lo dico ogni volta.

Senatrice Moronese, l'ho già detto, forse era distratta.

Tutto questo non fa parte - o meglio, non dovrebbe - della nostra decisione, che dev'essere basata sui fatti e sull'applicazione o meno della legge n. 1 del 1989.

uso la sua citazione in generale come pretesto per introdurre l'argomento caste e legge - perché stiamo parlando dell'applicazione di una legge che consente in assoluto, a chi svolge funzioni di Governo, di non andare a processo, se ricorrono determinate questioni. Su questo siamo riuniti oggi, poi il resto lo discutiamo tutti i giorni (la politica dell'immigrazione, giustizia e politica; temi che sono pane quotidiano). Quella del 1989, approvata in epoche lontane - non so neanche chi fosse fisicamente in Parlamento in quegli anni - non è una legge per favorire alcune caste, ma per consentire ad azioni di Governo di Governo di svolgersi, in presenza di determinati requisiti, senza impedire alla magistratura d'ipotizzare un'azione giudiziaria nei confronti di chicchessia al Governo, ma soltanto di sottoporre a una procedura

che vedo riemergere in questi giorni, con scampoli di dibattito e polemica. Infatti, è un problema ricorrente, con cui l'Italia e il mondo fanno i conti e i vari Governi - quali che siano le loro composizioni - si devono misurare, a volte cambiando opinioni,

che forse anche oggi trova un altro piccolo capitolo dell'uso politico da parte del Senato di una procedura giudiziaria. Resto convintissimo di quello che ho proposto all'Assemblea e mi auguro che il voto sarà favorevole. Ho ascoltato l'intervento del senatore Renzi, che ha posto un tema della giustizia e della politica. Questa è un'occasione per tutti, trasversalmente, per ribadire che un conto è governare un Paese e altro l'uso politico della giustizia: rinunciarvi è un grave errore

non il sovranismo dei comizi, ma la sovranità popolare, quella della Costituzione (perché la parola «sovranità» è scritta anche in Costituzione, non è una parolaccia).

Presidente, mi scuso per l'episodio precedente e capisco che era un momento di euforia, ma vorrei tranquillizzare la senatrice Moronese, dicendo che stavo cercando semplicemente di aprire una scatoletta di tonno. Tutto qua. *(Applausi.

mi ha ricordato i tempi in cui, da giovane militante di destra, mi opponevo anch'io a chi mi voleva impedire di parlare e manifestare le mie idee. giovani usavamo allora questa frase bellissima di Ezra Pound, che - sembra incredibile - dopo tanti anni è ancora attuale, perché c'è ancora chi pensa di chiudere la bocca a chi difende l'identità e la sovranità nazionali, come allora facevamo noi e come ha fatto lei da Ministro.

in particolare voterò a favore della relazione del presidente Gasparri, perché condivido appieno quanto ha detto il procuratore di Viterbo, dottor Paolo Auriemma, nel famoso colloquio con il dottor Palamara: «Non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il Ministro dell'interno interviene, perché questo non avvenga». Parole più chiare non potrebbero essere scritte. Palamara insiste, dicendo che va attaccato comunque e il procuratore di Viterbo replica: «Indagato per non aver permesso l'ingresso a soggetti invasori. Siamo indifendibili»,

Alcuni colleghi della maggioranza, prima, hanno insistito sul fatto che la nave Open Arms, come tante altre imbarcazioni delle ONG che navigano nel Mediterraneo, abbia operato soccorso in mare nei confronti di naufraghi. Invece siamo convinti che gran parte di queste navi e ONG non faccia soccorso in mare nei confronti di naufraghi, ma svolga un servizio di taxi del mare tra una sponda e l'altra del Mediterraneo, caso - molto spesso proprio laddove ci sono i barconi che improvvisamente non sono più in grado di navigare.

per soccorrere queste persone, che, come ho detto nella discussione generale, molto spesso, quasi sempre, non sono profughi né scappano dalla guerra, ma persone in cerca di fortuna e di migliori condizioni economiche, tra le quali molto spesso si annidano delinquenti o purtroppo anche persone che persone che diventeranno oggetto di sfruttamento (tra lavoro nero, prostituzione e quant'altro). Ebbene, siamo convinti che difendere i confini nazionali sia sempre e comunque un atto dovuto, che tutta la politica, destra e sinistra insieme, dovrebbe esercitare. Ho detto e ripeto che non mi meraviglio che da sinistra si voglia negare il perseguimento di un preminente interesse pubblico, laddove il Ministro abbia cercato di difendere i confini nazionali; da parte di chi nega il concetto stesso di identità nazionale e i confini e vorrebbe che non ci fossero confini e che tutti fossero liberi di andare dove vogliono e fare quello che vogliono, fregandosene della sicurezza

del Governo, condiviso ampiamente dal Presidente del Consiglio e dagli altri ministri interessati, che hanno emanato il decreto interdittivo del 1° agosto, in base al quale - ve lo ricordo - era vietato l'ingresso nelle acque territoriali italiane. Lo dobbiamo dire e ripetere a chi nega che ci fosse il perseguimento della difesa della legalità nell'operato del Ministro. Per tutte queste ragioni, cari colleghi, penso che oggi renderemo un servizio alla giustizia, affermando in questa sede che il Ministro ha operato nella funzione

Signor Presidente, colleghi, siamo di nuovo qui, per la terza volta, a decidere se autorizzare o no il processo nei confronti di Matteo Salvini per una questione relativa al sequestro di uomini, donne e bambini a bordo di una nave. fatti risalenti a un anno fa, quando il senatore era Ministro della Repubblica, incombenza dalla quale ha autonomamente deciso di sollevare se stesso, con sollievo di noi tutti e del Paese, in quegli stessi giorni di agosto. Possiamo dire che il caso Open Arms è il canto del cigno di un'esperienza ministeriale e di un certo modo di fare politica. Anch'io credo nelle mie idee e anch'io, come il mancato ministro Salvini,

sintetizzerò al massimo le questioni tecniche e giuridiche della vicenda che ciascuno di noi a questo punto conosce a menadito. È ormai chiaro a tutti il quadro normativo, nazionale e internazionale, di riferimento: l'obbligo di salvare la vita umana di chi si trovi in situazione di pericolo in mare prevale su ogni altra norma nazionale o accordo finalizzato al contrasto dell'immigrazione. Prevale, oltre che per una normale e ragionevole regola di civiltà, perché è un principio che, nella gerarchia delle fonti, ha un rango primario e dunque superiore. Chi difende Salvini parla di un'azione collegiale del Governo e di un preminente interesse pubblico. Come ho spiegato in Giunta e in discussione generale, non ci fu alcuna collegialità,

Mi dispiace che proprio in questo momento il senatore Gasparri abbia abbandonato l'Aula con il suo telefonino, perché vorrei ricordargli che probabilmente non ha seguito con attenzione il mio intervento, visto che cosa diversa è l'assistenza dei minori

quindi un intervento del presidente Conte c'è stato, è stato per ripristinare la legalità nazionale e internazionale, rispetto ad un'azione che era contro i minori e contro il diritto internazionale. quindi certamente un atto del Governo. Ciascuna azione di un Ministro deve però sempre e comunque svolgersi all'interno di una cornice di legalità costituzionale e internazionale, in modo che non si incorra nel pericolo che, in forza di una presunta ragion di Stato, vengano lesi diritti inviolabili dell'uomo, che pertanto sono ineludibili. Mi dispiace ripetermi, ma voglio anche oggi sottolineare che autorizzare il processo nei confronti del senatore Salvini è di estrema e delicata importanza. Dobbiamo infatti ribadire con forza il principio, negato da quest'Assemblea sulla vicenda Diciotti, per cui ciascuno è chiamato a rispondere alla legge quando decide deliberatamente di ignorarla, soprattutto per fini politici e di propaganda. Tale Tale convincimento - lo dico anche *pro futuro* - non è in alcun modo frutto di pregiudizio ideologico, come qualcuno ha affermato, nei confronti della persona. Al contrario, ciò che sostengo oggi che ho sostenuto nelle precedenti occasioni, lo sosterrò con la stessa forza in futuro, se mai dovessimo trovarci a prendere la stessa decisione su chi ricopre o ricoprirà la carica di Ministro dell'interno, perché le mie scelte si basano su considerazioni esclusivamente giuridiche e dovrebbe essere così anche per la Giunta, che è un organo di garanzia. Abbiamo invece visto che non è così: lo dimostrano i diversi risultati sulle tre autorizzazioni a procedere nei confronti di Salvini; lo dimostra la decisione incostituzionale sul seggio siciliano assegnato in Umbria; esiste però un caso, quello dei seggi della Campania, che fotografa l'inaccettabile atteggiamento che, senza distinzioni tra maggioranza e minoranza, attraversa la politica di questo periodo. La legge elettorale, che non ho condiviso nel merito e nel metodo di approvazione, definisce precisamente i meccanismi di assegnazione dei seggi. Il primo relatore di Forza Italia, senatore Malan, ha giustamente riconosciuto che il seggio spetta a Liberi e Uguali. Con una forzatura interpretativa della legge elettorale e della Costituzione, invece, si cerca da mesi, per ignote ragioni, di attribuire il seggio al ricorrente Lotito o magari confermare chi può vantare l'ultimo cambio di schieramento. Tornando alla Open Arms, è necessario fare alcune considerazioni: la prima riguarda i decreti Salvini, che sarebbe azzardato definire ancora decreti sicurezza, come vorrebbe il suo estensore. È evidente - e in quest'Aula l'ho già ribadito - che quelle norme sono esclusivamente propagandistiche e non hanno centrato l'obiettivo che si ponevano, ovvero sollevare l'*ex* ministro Salvini dalle conseguenze delle sue decisioni. Nel frattempo, la Corte costituzionale, una sentenza alla volta, li sta smantellando, sopperendo all'inerzia dell'attuale maggioranza. Invito i colleghi senatori che sostengono questo Governo a liberare da tale incombenza la suprema Corte e di procedere, senza ulteriore ritardo, alla cancellazione delle norme previste in tema d'immigrazione, se non per convinzione etica e giuridica, perché sono evidentemente dannose per una corretta gestione del fenomeno migratorio e non solo nell'ottica dell'integrazione, ma anche in quella della sicurezza. Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle: so bene che avete votato a favore di entrambi i decreti, ma è tempo di prendere atto dell'errore commesso e avviare un ravvedimento operoso che ripristini un impianto normativo degno di una democrazia compiuta, quale siamo. Lo dico anche ai colleghi del Partito Democratico, la cui linea sul tema comprende un ventaglio di posizioni fin troppo ampio. Lo dico ai colleghi di Italia Viva: al di là di quello che pensano gli intellettuali citati dal senatore Renzi, non dimentico che l'operazione Mare Nostrum fu cancellata dal suo Governo. Salvare le persone in mare è un obbligo: su questo non decidono il Governo o la maggioranza politica del momento; la gestione delle migrazioni invece sì, ha a che fare con la politica estera, con la sicurezza e con le scelte di politica economica e del lavoro, come quelle del *welfare*. ora - si deve cambiare. Questo è uno dei punti alla base della nostra fin qui leale e fin troppo paziente partecipazione a questa maggioranza. È un atto politico, la cui responsabilità non può e non deve ricadere ipocritamente sul solo ministro Lamorgese, perché riguarda il Governo nella sua interezza, tutte le forze politiche che ne fanno parte e ciascun deputato e senatore di maggioranza. Concludendo, abbiamo il dovere di ristabilire il principio di legalità, autorizzando il processo - badate bene: non la condanna, ma il processo - nei confronti del senatore Salvini. Non c'è sovranismo che possa prescindere dal rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali e delle leggi. Non c'è «prima gli italiani» che tenga, senza citare i diamanti in Tanzania, la laurea in Albania, la restituzione di fondi pubblici in comode rate ottantennali e i soldi in Svizzera. Abbiamo altresì il dovere politico e morale di superare gli accordi con la Guardia costiera libica, ai cui vertici abbiamo visto personaggi ambigui ed *ex* trafficanti, come il noto Bija. È di due giorni fa la notizia dei tre migranti uccisi e di altri feriti da membri della Guardia costiera, quando, non appena riportati a terra, hanno provato a fuggire, per non essere portati nei centri di detenzione. Mi pare evidente che rifinanziare la Guardia costiera libica sia tutto il contrario di quel che dobbiamo fare per risolvere il problema dell'immigrazione. Abbiamo il dovere politico di cancellare i decreti Salvini e chiudere definitivamente con una stagione fatta di propaganda, che continua, ora con meno successo, nella più totale irresponsabilità politica e istituzionale e abbraccia addirittura le teorie negazioniste del Covid-19. Abbiamo infine il dovere di stabilire, una volta per tutte, che Paese vogliamo essere e se siamo in grado o no di difendere e tramandare i valori scolpiti nei principi fondamentali della nostra Costituzione. Per tutte queste ragioni, dichiaro il voto contrario dei senatori della componente Liberi e Uguali alla relazione approvata dalla Giunta

Anna Rossomando, nel suo intervento, ha già spiegato ampiamente le ragioni di merito per cui voteremo contro la relazione della Giunta e ha già spiegato che il nostro compito, oggi, non è decidere se condannare o no Matteo Salvini per sequestro di persona plurimo o rifiuto di atti d'ufficio. Quello è un compito che spetta ai giudici, dobbiamo decidere se, nella vicenda della Open Arms, il Ministro dell'interno di allora abbia compiuto atti giustificati dal preminente interesse pubblico o no. Per noi la risposta è no, perché non è credibile l'argomento usato, anche nella relazione del presidente Gasparri, ossia la presenza a bordo di terroristi. Se fosse stato così, perché dopo un anno nulla è successo e non ci sono stati un arresto o un'indagine che abbia portato a qualcosa? Perché? Dove si evidenziava questo pericolo? Per noi non è neanche dimostrato - ammesso che ciò potesse giustificare la scelta di lasciare in mare 160 persone per diciannove - né dimostrabile che ci fosse la necessità di fare pressione sull'Europa per la ripartizione di quelle persone; anzi, è dimostrato che la disponibilità ad accogliere, da parte di diversi Paesi europei, era già stata ottenuta dal Presidente del Consiglio. non è dimostrato l'interesse pubblico, ma, anche se lo fosse, voglio dire con grande chiarezza che non pensiamo che esso possa giustificare le violazioni dei diritti umani e delle libertà individuali e le sofferenze di quelle persone,

possibilità di giustificare quello che è successo. Non esiste un interesse pubblico che possa giustificare quelle violazioni e la scelta di non prendersi cura di persone in difficoltà. Questo non c'entra niente con il controllo dei confini e dell'immigrazione, o la necessità di sollecitare un impegno maggiore dell'Europa: non c'entra nulla! C'entra forse con la propaganda e con il bisogno di mostrare come vera la tesi della chiusura dei porti e di nascondere l'inutilità di politiche che mostravano di accanirsi sui migranti e non sugli scafisti. Il fine giustifica i mezzi. Se mostriamo la faccia cattiva del Paese, nessuno partirà più. Inutilità che si voleva nascondere dimostrando durezza e intransigenza nei confronti di uomini e donne salvati dal mare, a cui sono stati riservati trattamenti disumani. Nascondere il fallimento di quelle politiche: questa era la finalità di quell'atto.

ossia che mentre teneva in ostaggio 160 persone al largo di Lampedusa, negli stessi momenti, centinaia di persone, ogni giorno, arrivavano lì e sulle nostre coste dalla Tunisia, semplicemente perché quel

e sta succedendo quello che è successo un anno fa, con la differenza che il ministro Lamorgese, per fermare questi flussi, è andato in Tunisia e ha aumentato la presenza delle Forze dell'ordine in Sicilia, mentre un anno fa si negava l'esistenza del problema, che bastasse tenere Open Arms in mare per diciannove giorni, per dimostrare di saper contrastare l'immigrazione. Altro che interesse pubblico: il rischio vero è quello di fare propaganda sulla pelle delle persone salvate. ripeto che non spetta noi dire o decidere se il senatore Salvini è colpevole o innocente; a noi spetta il compito di consentire alla magistratura di decidere, perché nessuno è al di sopra della legge e uno Stato democratico e garantista non può non valutare fino in fondo se l'equilibrio tra interesse pubblico e diritti individuali è stato oltrepassato o meno. Se il senatore Salvini è convinto delle sue ragioni, come dice, penso che, come l'ultima volta, dovrebbe rimettersi al giudizio di un tribunale.

che il senatore Salvini venga condannato; non siamo quelli del buttare via le chiavi, delle manette facili, o del mettere la gente in carcere per qualsiasi cosa. Ci auguriamo che il senatore Salvini venga assolto, ma continueremo a combattere la sua idea di Paese e la sua politica forte con i deboli, che vuole agitare i problemi anziché risolverli. Guardi, senatore Salvini, non c'è alcuna via giudiziaria che vogliamo seguire. Non siamo come lei: non facciamo giustizia sommaria; non usiamo le inchieste come lei fa ogni volta che può. Ci siamo dimenticati di Bibbiano, e dell'Umbria e dell'Umbria e di come viene strumentalizzata ogni notizia di reato che riguarda una parte diversa dalla propria? *(Applausi)*. Chiediamo solo che si faccia chiarezza e si possano esprimere i giudici per rispetto della magistratura.

si è convertita al garantismo, ma lo ha fatto a seconda delle situazioni, solo quando conviene. Si erge a censore di fronte a ogni notizia di reato o sospetto che riguarda gli altri e poi non sente mai il bisogno di chiarire vicende che chi vuole governare la cosa pubblica dovrebbe chiarire. Si chiamino i 49 milioni (dove sono?), si parli dei fondi dalla Russia, si parli dei camici, si parli dei paradisi fiscali. Non se la può cavare; nessuno se la può cavare con la teoria del complotto. Bisogna rispettare i cittadini. Le gravissime cose che emergono dalle intercettazioni di Palamara vanno certamente perseguite. Servono riforme e le stiamo facendo; ma nessuno può usarle per delegittimare la magistratura o, meglio, per difendere se stesso. I magistrati che fanno le indagini che non piacciono, sono sempre loro quelli che vengono messi in croce. E non può neanche usarle per non rispondere mai a ciò che riguarda lei, senatore Salvini, o il suo partito. Io credo, senatore Salvini, che lei

trattandoli con disprezzo e con dispregio. *(Applausi)*. Invece di raccontare di tutto, meno che delle cose di cui deve rispondere, farebbe meglio oggi a dare risposte agli italiani sulle questioni che riguardano lei, anche su questa questione, e a dare spiegazioni che capiscano anche i bambini di sei anni, a cui spesso si rivolge. Stia tranquilla anche la senatrice Stefani: non abbiamo scelto nessuna via giudiziaria. Noi vogliamo battervi politicamente, dimostrando che anche i grandi problemi come quello dell'immigrazione possono essere governati senza mai perdere di vista i diritti e le libertà delle persone, semplicemente continuando a essere umani.

Signor Presidente, mi sembra di rivivere un'esperienza che abbiamo vissuto insieme nel 2013, quando, come oggi, una parte di questo Senato, ignorando e violando la legge, applicò una sanzione sbagliata al presidente Berlusconi. Violando la legge! *(Applausi)*. Non lo dico io: l'ha detto la Corte di cassazione a sezioni unite nel giugno 2019. Avevate detto che non potevate valutare le questioni di costituzionalità, perché la Giunta delle elezioni era un organo paragiurisdizionale la Giunta delle elezioni era un organo paragiurisdizionale e il presidente Grasso consentì la votazione palese su queste questioni. Sappiamo benissimo che le sezioni unite della Corte di cassazione hanno detto che è un organo giurisdizionale di natura costituzionale. Non solo. Nella stessa vicenda, voi sapete bene che diceste che non si può discutere la sentenza della Cassazione. Sapevamo tutti che era sbagliata. Lo dico io? No, la Corte di cassazione, otto mesi dopo, nel marzo 2014. Quella sentenza non poteva essere applicata perché non aveva alcun principio di diritto.

senatore Mirabelli, non è vero che voi volete rimettere la questione alla magistratura; non c'entra nulla. Non giudicando oggi voi quello che vi spetta di giudicare, non potrà essere giudicato da nessuno. La legge costituzionale del 1989 dice che spetta al Senato quella valutazione, non alla magistratura. La magistratura non potrà valutare se sussiste o meno un interesse pubblico.

Perché il legislatore costituzionale ha attribuito al Senato e non al giudice la valutazione di una esimente, di una causa di giustificazione come tutte le altre? L'adempimento del dovere è già previsto ed è quello che viene giudicato dal giudice ordinario. Qua invece è la norma costituzionale. Ho sentito alcune letture di sentenze della Corte di cassazione sbagliate, perché la lettura che si faceva della sentenza della Corte di cassazione si riferisce alla questione della tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante. Questa esimente, la relazione del senatore Gasparri non la prende in considerazione e dice correttamente prende, invece, in considerazione l'altra esimente, ovvero il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

legittima difesa putativa. Sul perseguimento dell'interesse pubblico si tratta di valutare qual è l'interesse pubblico: un programma di Governo è un interesse pubblico o no?

abbiamo votato una proroga dello stato di emergenza sanitaria. Secondo lei, è possibile individuare un interesse pubblico nel mantenimento delle elezioni al 20 settembre o del voto su una riforma costituzionale? No, vi è una contraddizione in termini. In democrazia, se c'è un'emergenza sanitaria non si fanno elezioni, in qualsiasi Paese al mondo. mondo. La vera democrazia è nel momento elettorale, quando la gente può partecipare, discutere, ragionare e partecipare al dibattito politico-amministrativo, ma tutto ciò non sarà possibile.

bisognava individuare una legge che consentisse l'ingresso legale nel nostro Paese; bisognava salvare le norme che riguardavano il diritto asilo e i rifugiati, ma bisognava pur stabilire delle regole che non consentissero l'ingresso di tutto il mondo nel nostro Paese e che, oltre i limiti fissati dall'ingresso legale, non era possibile accogliere tutti.

il senatore Salvini e sappiamo tutti che in quei quindici giorni tutti sono stati coinvolti, ma non l'Italia. Quindi dite una bugia.

Palamara e Auriemma erano d'accordo che Salvini non c'entrasse; la loro valutazione era che Salvini fosse innocente che non si potesse applicare quella legge. Ma si diceva: "Però diamogli addosso". E questa è la logica con cui state ragionando. ragionando. O mi identificate un qualcosa che doveva essere fatto e che non è stato fatto, oppure, se fossi il giudice - non sono l'avvocato, ma non sono nemmeno il giudice dovrei interrogarmi sul perché davanti a me si trova soltanto Salvini e non Conte, e non gli altri Ministri che hanno firmato con Salvini. noi ci troviamo di fronte non a questa attività. Noi esercitiamo una funzione propria, quella del componente del Senato che deve valutare se esista o meno una esimente che non può valutare nessun altro. E la causa di giustificazione esiste o no? Sì, perché vi è un interesse pubblico. Come fate a dire che non c'è un interesse pubblico una volta che sono state approvate delle leggi che vincolano tutti, che devono garantire i flussi migratori e la sicurezza del nostro Paese. Tant'è vero che il presidente Grasso, con la sua bravura, per tentare di annacquare ha detto che vi era un generico rischio di terrorismo. Presidente Grasso, lei ricorda, come me, gli anni Settanta, quando si parlava di sedicenti Brigate Rosse. E dopo qualche anno ci siamo trovati con i morti per la strada. Allora il generico rischio del terrorismo non era un generico rischio; sappiamo tutti che cosa avviene che cosa ci portano nel nostro Paese. *(Applausi).* Quando vi è un flusso migratorio non regolato e non controllato, abbiamo queste conseguenze. Come fate a voler violare la legge? Perché la vostra decisione sarebbe contro la norma. E chi la interpreta, allora? Non lo potrà fare il giudice, perché questa è una funzione nostra. E chi si rifiuta di farlo, viene meno alla propria funzione. Voi state mettendo in atto una attività che è contro la funzione del senatore, perché non avete diritto né avete la necessità

Oggi, come fa a non prendere in considerazione l'interesse pubblico che era frutto di leggi approvate da voi, non da me? Io oggi ho chiesto di intervenire alla presidente Bernini - e la ringrazio - semplicemente per affermare dei princìpi, delle regole. Poi mi interessa meno se si tratti di Salvini o di altri. Mi interessa il rispetto delle regole che il Senato deve avere perché, nel momento in cui questo non si realizzasse, ci troveremmo di fronte all'anarchia più totale, alla democrazia che calpesta se stessa. Nel momento in cui le norme non trovano applicazione nel luogo e nel tempo in cui devono essere applicate, è la negazione dello Stato democratico. E su questo credo che ciascuno di noi debba interrogarsi.

Signor Presidente, senatrici e senatori, iniziamo con una domanda: come mai ci sono state queste tre domande di autorizzazione a procedere su fatti palesemente collegiali, e in tutte e tre le domande si chiede solo di processare Salvini? *(Applausi).* Nel caso Diciotti - non so se qualcuno lo ricorda

Negli altri due casi non ci sono state analoghe memorie, ma ci sono ampie dichiarazioni pubbliche, che ho richiamato anche nel precedente intervento. Eppure, nulla. Non ho una risposta tecnica, da penalista, perché il concorso nel reato c'è ogniqualvolta più persone condividono, a prescindere dal ruolo che ciascuno ha. allora un'altra domanda. Poco fa Salvini diceva: «Lo so, qui ormai avete deciso di votare contro di me». allora quale sarebbe stato l'esito del voto oggi, se la domanda di autorizzazione a procedere, oltre che Salvini, avesse incluso anche Conte e gli altri Ministri competenti.

dunque queste parole e ogni parola ha un senso. Prima dice: «Hai ragione», quindi io Palamara reputo che è vero che Salvini interviene affinché non ci siano ingressi illegittimi, è vero che sta facendo il suo dovere (e forse è anche vero: cosa c'entra la procura di Agrigento?),

«noi magistrati» non è che «possiamo attaccarlo», ma «dobbiamo attaccarlo», anche se sta dalla parte della ragione.

«Indovina chi è il presidente del tribunale dei Ministri di Palermo? Io!»: cioè, questa guerra dichiarata a Salvini era talmente nota, quantomeno tra i magistrati, da indurre indurre chiunque si trovasse ad avere un fascicolo in mano riguardante Salvini a scrivere immediatamente a Palamara. «Lo sai chi se ne occupa? È stranissima una cosa del genere. E sapete cosa risponde Palamara, sempre sobrio, discreto, che tutela le istituzioni? Risponde: «Grande». Grande, e poi conclude, dopo la chiacchierata: «Io «Io sono sempre con te. Un abbraccio forte». Considerate che quasi tutte le *chat* di Palamara si concludono con un abbraccio: qui forse era una figura particolarmente importante e in quel momento l'abbraccio è «forte». Quando sono venuti alla luce questi messaggi, per due o tre giorni tutti si sono scandalizzati sui giornali e poi si è detto: tutto sommato c'è un processo a Perugia, vedremo cosa succederà. Il processo di Perugia, per chiarezza, verificherà se gli eventuali reati a carico di Palamara sussistono. Ma io mi pongo un altro problema: se quelle non erano chiacchiere private (perché non mi sembrano chiacchiere private, visto che tutti sapevano qual era l'obiettivo di Palamara), questo invito di Palamara è rimasto soltanto in quella *chat* o, per caso, ha avuto conseguenze? Vediamo un po' di date? Lo sapete di che data è quel messaggio? Agosto 2018.

qualsiasi tipo di ritardo o di diniego allo sbarco illegittimo si trasforma in sequestro: Diciotti, sequestro; Gregoretti, sequestro; Open Arms, sequestro. Si dirà: forse è perché, alla fin fine, Salvini comincia a operare in quel momento, quindi effettivamente è da quel momento che si configura un reato. La risposta è: mi dispiace, ma non è così, perché le stesse identiche condotte, ritardo o diniego, si verificano anche successivamente, senza conseguenze penali: ottobre 2019, Governo Conte è caratterizzato da porti spalancati, ma non sempre. L'Ocean Viking viene bloccata in mare per undici giorni

uno era un presunto sequestro per tutelare la Patria e l'altro era un sequestro per fini elettorali. Ma, attenzione, io noto due pesi e due misure anche su un altro fronte: sapete chi è Creus? È un personaggio importante, a volte fa anche interviste con Baricco e altri.

altri viaggi fatti da Open Arms in passato. Cosa succede a Creus? Nel marzo 2018 era per caso ministro Salvini? No. Ebbene, Open Arms, con il comandante Creus, fa il solito giochino di chiedere con insistenza di arrivare in Italia; sbarca in Italia e scatta un processo a suo carico per reati gravissimi.

perché anziché dirigersi verso Malta, punto di sbarco più vicino, e richiedere alle autorità maltesi l'indicazione di un porto, così come previsto dalle convenzioni internazionali e come indicato dallo Stato di bandiera, si dirigeva verso le coste italiane, costringendo le autorità italiane

Cosa succede al Creus delinquente? Delinquente secondo quella richiesta di rinvio a giudizio, Creus è a bordo della Open Arms nell'agosto 2019, Salvini vi ha già ricordato che Creus, per quattro volte, rifiuta la possibilità di far sbarcare i migranti. Vediamo quali sono queste

non fa scendere i migranti. Il 18 agosto, primo benestare spagnolo e la risposta di Creus è la seguente: troppo lontano arrivare fino allo Stretto di Gibilterra.

Il 19 agosto, per eliminare ulteriori alibi, si indica un porto ancora più vicino, Gibilterra. Creus rifiuta per la quarta volta. Allora, la mia domanda è: se c'è una situazione di pericolo, e tu hai la possibilità, per quattro volte di uscire dalla situazione di pericolo e dici di no, tu, sei uno che se la va a cercare o no?

non ha imputazioni. Sapete chi ha l'imputazione di rifiuto? Matteo Salvini. Perché, oltre al sequestro, ti segnalo, Matteo, che ti hanno dato anche il rifiuto di atti d'ufficio. Quello rifiutava, ma il reato lo davano a lui, che è il re Mida del reato: dove tocca, è reato.

quali aperte e una chiusa, blindata, e io, anziché dirigermi serenamente verso le quattro porte aperte, cercassi di forzare quella chiusa, sarei vittima di un sequestro oppure sarei una pazza scatenata che cerca in tutti i modi di forzare una porta? *(Applausi).*

che ci sono situazioni diverse e che non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio, ma è anche vero che, tra alcune di queste navi, mi sembra che si stiano iniziando a fare un po' di capricci: lì non vado, lì neanche, neanche lì; quindi,

forse si deve anche tener conto del fatto che c'è un interesse pubblico anche ad evitare che soggetti che hanno accuse pesantissime, come quella di favoreggiamento, entrino in Italia. Ve lo siete posti questo problema? Vorrei dire un'altra cosa. Voi che adesso vi accingete a votare per mandare a processo Salvini, siete a favore di Creus. Vorrei segnalarvi un fatto che forse vi è sfuggito. Sapete cosa è successo il 5 febbraio 2020? A Ragusa è iniziato il processo a carico di Creus. Chi oggi vota contro Salvini dice che Creus è perbene. Bene, chi sostiene questo Esecutivo sappia che il Governo si è costituito parte civile contro Creus il 5 febbraio scorso. *(Applausi)*. Sapete chi si è costituito parte civile?

dell'interno. Il giudizio sulla politica dell'immigrazione del ministro Salvini verrà definitivamente sottratto alla valutazione della storia e dell'elettorato e lo affiderete alla magistratura.

attacca Salvini pur sapendo che ha fatto il suo dovere. Siete dei parlamentari, non inginocchiatevi a Palamara!

in quest'Aula il senatore Matteo Salvini ha affermato testualmente che i porti aperti hanno salvato vite, i porti chiusi condannano a morte migliaia di persone. Possiamo chiederle, collega Salvini, se si è trattato di un ravvedimento? Credo, più probabilmente, a un *lapsus* - purtroppo - perché, in realtà, nell'agosto 2019 l'ex ministro Salvini privava della loro libertà personale 161 naufraghi, poi diventati 134 (tra (tra cui un neonato di nove mesi, due bimbi e due donne in gravidanza), stipati in una nave civile che poteva contenere al massimo 19 persone, sotto il sole, privi di dignità umana, reduci da guerre, sofferenze, violenze e da un naufragio; persone persone psicologicamente stremate e malate, come provano le numerose evacuazioni mediche che vennero disposte. Ricordiamo anche che a bordo della nave, nei giorni a cavallo di Ferragosto, la situazione sanitaria andava peggiorando di ora in ora, con alcune persone che giacevano in condizioni molto serie, con carenza di antibiotici e in presenza di infezioni da arma da fuoco. Alcuni migranti, alla vista della terraferma, decisero di lanciarsi in mare nel tentativo di raggiungere la costa a nuoto per circa 800 metri. Ex ministro Salvini, parliamo di persone che furono fatte sbarcare solo dopo venti giorni e non da lei, ma dalla Procura di Agrigento. mentre sulla nave si consumava questo dramma, il senatore Salvini cavalcava le scene sui palchi, convinto di essere già in campagna elettorale per le politiche, affermando, in maniera rozza e disumana, che era finita la pacchia per chi voleva sbarcare in Italia.

per i reati di sequestro di persona aggravato e violazione di doveri d'ufficio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Occorre pertanto chiedersi: Salvini agì nell'ambito di un'azione governativa allo scopo di perseguire un preminente interesse pubblico, come richiede la scriminante di cui all'articolo 9 della citata legge, oppure da solo e per un suo personale convincimento politico? Ebbene, il Gruppo MoVimento 5 Stelle oggi c'è, è presente e non ha dubbi. L'allora ministro dell'interno Matteo Salvini, con un grave comportamento assunto autonomamente e non condiviso dalla restante compagine governativa, in aperta violazione delle norme di diritto internazionale e dei princìpi di rango gerarchico superiore che impongono agli Stati firmatari l'obbligo di salvare le vite in mare, trattenne illegittimamente le persone a bordo, negando loro lo sbarco per un suo convincimento politico che non può assurgere a preminente interesse pubblico dello Stato e dei suoi cittadini e per questa ragione dovrà essere sottoposto a procedimento penale davanti all'autorità giudiziaria. Lasciamo alla magistratura ogni valutazione e non facciamo in questa sede nessuna condanna. Pertanto il MoVimento 5 Stelle esprime dissenso rispetto al pronunciamento della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ha accolto la proposta del presidente Gasparri di negare l'autorizzazione a procedere. Ciò non senza rilevare che la proposta citata, in particolare in sede di replica alle numerose eccezioni sollevate anche dal MoVimento 5 Stelle in Giunta, contiene una vistosa forzatura interpretativa, direi quasi ermeneutica, dei fatti e della loro cronologia. Innanzitutto il relatore richiama nei suoi scritti solo parzialmente le note scritte del *premier* Conte e si è spinto a sostenere che solo con la lettera del 16 agosto, indirizzata all'allora Ministro, il presidente del Consiglio Conte avesse esplicitato la linea da seguire, ma così non è. Già nella prima missiva, quella del 14 agosto, infatti, il Presidente del Consiglio indicò in modo chiaro la linea da adottare per risolvere quello che nel frattempo era divenuto il caso Open Arms, sollecitando Salvini - queste le sue parole - ad adottare con urgenza i necessari provvedimenti per assicurare assistenza Grazie a tutti che impone agli Stati firmatari, tra i quali l'Italia, l'obbligo di soccorrere e prestare assistenza alle persone in mare, ma soprattutto l'obbligo di portare queste persone in un luogo sicuro e quindi sulla terraferma.

(frasi affermate da Salvini da un palco durante un comizio). Ci si chiede tuttavia che importanza poteva avere la circostanza che di 27 soggetti minori, in realtà nove risultarono maggiorenni: evidentemente nessuna. Così però non è stato per la maggioranza dei componenti della Giunta e per il presidente Gasparri, i quali invece sostengono, davvero arditamente e in spregio alla reale successione dei fatti, che l'indirizzo dato dal presidente del all'allora Ministro sia datato 16 agosto invece del 14, quando il Presidente del Consiglio richiamava espressamente Salvini al rispetto della normativa in vigore. A ciò si aggiunga che i minori, dopo l'ordine di Conte e l'intervento del tribunale per i minorenni di Palermo, vennero fatti sbarcare solo il 17 agosto da Salvini, suo malgrado (sono state le parole dell'ex Ministro). Non è vero, quindi, lo sbarco avvenne immediatamente o lo stesso giorno della presa d'atto da parte di Salvini dell'indirizzo governativo, rispetto al quale invece ribadì la sua difformità per il suo orientamento politico.

presidente Gasparri ha scritto nella sua relazione iniziale, il diritto interno cede sempre il passo alle norme di diritto internazionale che prevalgono e non c'è bisogno di nessun ricorso alla Corte costituzionale. A nulla valse, peraltro, il tentativo disperato, fallito clamorosamente, del quale non si fa nessuna menzione nel provvedimento della Giunta, col quale Salvini, dopo che il TAR aveva sospeso il decreto sicurezza *bis,* cercò di emettere un altro provvedimento interdittivo, che però il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si rifiutarono di controfirmare, dando così quella prova inconfutabile che andate continuamente a cercare dell'aperto dissenso tra la linea adottata dall'ex ministro Salvini e l'indirizzo collettivo del Governo. Non possiamo neanche accettare un'altra temeraria e ardita deduzione fatta dal relatore, ossia che l'indirizzo dato dal Presidente del Consiglio riguardasse solo i minori. Aveva infatti chiarito in poche righe, il *premier* Conte, di aver ricevuto la disponibilità da parte di una pluralità di Stati all'accoglienza dei migranti della Open Arms, secondo le sue parole: «a condividere gli oneri dell'ospitalità per tutte le persone di cui ci stiamo occupando, anche indipendentemente dalla loro età». A nulla vale il parallelismo, anch'esso super sfruttato, tra il caso Diciotti del 2018 e i casi Gregoretti e Open Arms del 2019, casi concreti completamente diversi, per cui diverse devono essere le conclusioni. Nei mesi trascorsi tra le due estati, un pregevole lavoro diplomatico era stato portato avanti dal *premier* Conte, che aveva consolidato i buoni rapporti con i *partner* europei e la redistribuzione dei migranti era divenuta una buona pratica, che sarà infatti formalizzata ad ottobre, nell'incontro di Malta, sicché la pressione da fare sui Paesi europei tramite il divieto di sbarco dei naufraghi non era più un'azione governativa, ma l'azione politica assolutamente personale del senatore Salvini. ancora più singolare appare quindi l'argomentazione del presidente Gasparri, secondo cui non è necessario che il preminente interesse pubblico sussista veramente, ma sarebbe sufficiente la ventilata volontà del Ministro di perseguirlo. In questo modo, si giustificherebbe pienamente l'operato di Salvini, il quale sostiene di aver agito per scongiurare la minaccia terroristica legata ai flussi migratori, messa in evidenza durante una riunione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica tenutasi un anno prima, nel 2018. Questa altro non è che una scappatoia, frutto di una forzatura inaccettabile, che non tiene conto del profondo mutamento del panorama internazionale avvenuto nel 2019, allorché gli Stati europei decidevano di adottare la politica della redistribuzione, come inaccettabile è che si affermi che si deve apprezzare il fatto che Salvini volesse salvare l'Italia e gli italiani dal terrorismo internazionale, anche se questo rischio era del tutto immaginario. Accettare questa argomentazione significherebbe sovvertire un parametro oggettivo di giudizio e la logica stessa del giudicare, perché si finirebbe per dare giustificazione a qualsiasi azione criminale, se astrattamente finalizzata a perseguire un imprecisato interesse preminente, sganciato dalla reale portata dei fatti. Ultima, ma non meno importante annotazione, che dimostra come le idee del ministro Salvini e del Governo cui allora apparteneva fossero ormai su binari diversi e lontani: nei giorni della vicenda della Open Arms, si era consumata l'insanabile frattura voluta dallo stesso senatore Grazie a tutti una brutta pagina della storia repubblicana, macchiata ulteriormente dal tentativo strumentale e autoreferenziale della Lega di opporsi alla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del loro *leader.* È per tutti questi motivi che, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, dichiaro il voto contrario alla relazione del senatore Gasparri.

Signor Presidente, nei pochi minuti a mia disposizione vorrei parlare di due problemi. Il primo si chiama Matteo Salvini è diventato un simbolo. Il senatore Salvini è intervenuto spesso in quest'Aula ultimamente. Io faccio parte del suo schieramento ma non sempre mi sono trovato d'accordo con lui, anzi spesso le mie opinioni sono differenti. Ciò non toglie che, quando una persona diventa un simbolo, è un grave problema per la politica e addirittura un crimine per la giustizia. Questo bisogna in qualche modo tenerlo presente e avere un principio di precauzione ancora più forte. Signor Presidente, lei sa che non siamo nuovi in quest'Aula e sa che che questo principio di precauzione lo abbiamo avuto non solo quando si è trattato di prendere posizione nei confronti di persone del nostro schieramento, ma anche e soprattutto quando si è trattato di nostri avversari politici. Il secondo problema si chiama politica, signor Presidente, e in particolare si chiama *gubernaculum*: quello spazio di governo la cui difesa ha coinciso con la nascita del moderno costituzionalismo. Noi siamo qui a difendere l'imperio; la possibilità che non sia un altro potere, senza contrappesi adeguati, a decidere cos'è il preminente interesse pubblico. A me pare che oggi stiamo delegando questo potere alla magistratura. Sottrarre decisioni come quelle sul processare un Ministro alle dinamiche della post-politica è fondamentale se vogliamo ancora affermare un ruolo per questo Parlamento. La si può pensare come si vuole, come si vuole, si può cambiare una maggioranza, ma almeno quei senatori che facevano parte della precedente maggioranza non dovrebbero cambiare idea sull'interesse pubblico, altrimenti muore la politica e nasce la post- politica. Questo per decenza, ma se la decenza è morta noi vorremmo cercare di evitare che muoia anche la politica, ed è per questa ragione

dunque alla votazione. Ricordo che la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento, si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 160 voti. Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Matteo Salvini nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore*. I senatori favorevoli alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere voteranno sì. I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

che il risultato non verrà proclamato immediatamente. I senatori che non abbiano partecipato al voto potranno successivamente recarsi al banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alla chiusura delle operazioni di voto prevista per le ore 18. Successivamente si procederà allo scrutinio e alla proclamazione del risultato. La seduta non è sospesa. Alle ore 15 è previsto il *question time*.

Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, le misure restrittive alle attività economiche e produttive e sociali adottate per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno avuto quale conseguenza la crisi economica peggiore dal dopoguerra ad oggi. In particolare, tra i settori più colpiti c'è il canale Horeca(*hotellerie, restaurant, café*), cioè l'insieme degli operatori che lavorano nel settore della somministrazione degli alimenti e delle bevande, diversi dalla grande distribuzione organizzata che interessa prevalentemente il commercio del *food* e del *beverage.* Questo specifico comparto ha subito, da prima, la completa chiusura durante il *lockdown* e, successivamente, una complessa fase di riapertura con limitazioni dei posti a sedere legate alle necessarie misure di distanziamento sociale. Considerato che anche il flusso turistico ha registrato un calo senza precedenti e la pandemia non accenna a diminuire, in particolare fuori dai confini europei, la crisi del settore della ristorazione si sta ulteriormente aggravando. agricolo alimentare) sul fronte del consumo alimentare extradomestico, la spesa delle famiglie italiane, nel 2019, ha sfiorato gli 86 miliardi di euro, con un incremento reale sull'anno precedente dell'1,6 a fronte di tale andamento decisamente positivo, le prospettive dei consumi extradomestici per tutto il 2020 sono tutt'altro che incoraggianti: si può stimare prudenzialmente per il canale Ho.Re.Ca un calo pari al 40 per cento, per un ammontare che si aggirerebbe attorno ai 34 miliardi di euro di perdita; secondo "#FareRete", progetto composto da 30 associazioni del settore ristorazione con 100.000 addetti e secondo i settori agroalimentare e pesca dell'associazione "Alleanza delle cooperative in assenza del canale della ristorazione una quota compresa tra il 30 e il 50 per cento delle produzioni agroalimentari si trova priva di sbocco commerciale; secondo Coldiretti, solo nei 3 mesi di *lockdown* il crollo delle attività di ristorazione per il fermo forzato di alberghi, bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha avuto un effetto negativo che si è riverberato sull'intero settore agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di almeno 1,5 miliardi di euro per i mancati acquisti in cibi e bevande; le misure di liquidità e di aiuto a fondo perduto, introdotte con il decreto-legge "cura Italia" e con il successivo "decreto rilancio", sono state un primo segnale positivo ma non decisivo per risollevare il settore in questo contesto, aumenta il rischio di spreco alimentare legato alla mancata collocazione sul mercato delle produzioni destinate al settore della ristorazione, si chiede di sapere quali misure urgenti il Ministro in indirizzo stia elaborando per il sostegno diretto alle 180.000 attività di ristorazione e a beneficio dell'intera filiera agroalimentare italiana,

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emergenza Covid-19 e la prolungata chiusura di gran parte degli esercizi del settore Horeca hanno determinato perdite per tutti i soggetti economici coinvolti nel sistema agroalimentare. Anche la riapertura, in queste settimane, vive criticità che non possono essere ignorate, a partire dalla drastica diminuzione dei posti a disposizione nei locali, che si ripercuote sui fatturati delle imprese di ristorazione già in forte sofferenza e anche sui livelli occupazionali. In questi ultimi tempi, tutti abbiamo riconosciuto il ruolo strategico e determinante della nostra filiera agroalimentare, quella che abbiamo chiamato filiera della vita. Tutti abbiamo detto grazie, ma non basta. Sostenere la ristorazione significa impedire il venir meno di un pezzo strategico del nostro *made in Italy*, un pezzo su cui si fonda la nostra forza, la nostra identità nel mondo. Come ho già ribadito ai colleghi di Governo, la filiera agroalimentare italiana deve essere considerata nella sua prospettiva più ampia, dal lavoratore agricolo al consumatore. In quest'ottica, il settore della ristorazione rappresenta un anello cruciale, direi determinante, considerata soprattutto la quota significativa di prodotto agroalimentare nazionale, inclusi vini e bevande, che viene assorbita da ristorazione e pizzerie e che influisce in modo rilevante sui segmenti di eccellenza delle nostre produzioni. Con il ministro Patuanelli abbiamo ascoltato le rappresentanze del settore ed è quanto mai urgente intervenire per sostenere i ristoratori e la filiera tutta, nell'ambito delle azioni da prevedere nel prossimo decreto di sostegno ai settori economici e produttivi. In queste ore è in corso un'intensa attività di confronto con le altre amministrazioni, al fine di definire le modalità di intervento. La nostra proposta è già sul tavolo: un fondo per la ristorazione del valore complessivo di circa un miliardo di euro. È infatti necessario favorire il più possibile la fase di mantenimento in vita degli esercizi di ristorazione con una misura immediata che inietti liquidità per poter mettere queste imprese nelle condizioni di riattivare rapidamente le forniture di alimenti e che potenzi quanto già previsto nei decreti liquidità e rilancio. Da qui la proposta di un fondo *ad hoc* per un *bonus* filiera Italia. Proponiamo infatti un *bonus* di circa 5.000 euro a fondo perduto diretto ai 180.000 esercizi pubblici di ristorazione per l'acquisto di prodotti agroalimentari nazionali e da materie prime italiane. Come dicevo, l'obiettivo di questa proposta è duplice: garantire un'immediata iniezione di liquidità e sostenere, allo stesso tempo, la filiera agroalimentare italiana. Sono convinta che l'adozione di una misura di questa portata potrà contribuire in modo molto significativo a riattivare dinamiche economiche e sociali virtuose di cui il Paese, soprattutto in questo momento, ha profondo bisogno.

I nostri ristoratori sono il fiore all'occhiello del *made in Italy*, l'eccellenza della filiera enogastronomica. Da sindaco posso testimoniare la sofferenza, il disagio, ed anche il dolore alcune volte, di generazioni di famiglie che hanno tramandato un antico mestiere, che mai andrebbe deriso e abbandonato perché è uno dei collanti più importanti delle nostre comunità.

prevalentemente proveniente dal Canada. Parliamo di milioni di quintali, quantitativi non indifferenti che vengono destinati alle grandi aziende industriali alimentari, che alterano così anche i listini prezzi del mercato nazionale. Ufficialmente, sembrerebbe non sufficiente la quantità prodotta in Italia ma in realtà è proprio la situazione di mercato precaria che scoraggia la coltivazione di questo importante cereale per la nostra dieta mediterranea. Ricordo al Ministro che ho presentato molte interrogazioni, nelle quali ho riportato in maniera dettagliata tutti i dati delle navi, ma nessuna di queste ha ricevuto risposta, neanche in ordine ai controlli dell'Ispettorato centrale della tutela Informo il Ministro che il 27 luglio ha fatto visita proprio al gruppo Casillo che risulta essere il principale importatore di grano estero canadese. Infatti da inizio anno ha importato circa 1.650.000 quintali su un totale di oltre tre milioni di quintali che tutta l'Italia ha importato dall'estero. Vorrei anche ricordare al Ministro che in quest'Aula è stata approvata la mozione sul glifosato che è una sostanza presente nel grano canadese dannosa per la salute pubblica. Recenti studi scientifici ne hanno infatti messo in evidenza genotossicità, interferenza endocrina e alterazione del microbiota intestinale oltre alla probabile cancerogenicità. allora oggi al ministro Bellanova: quali iniziative intende assumere al fine di scoraggiare l'acquisto di grani esteri che vengono puntualmente miscelati con il grano duro nazionale di ottima qualità, deprimendone la produzione nazionale? Visto che lunedì il Ministro è stato a Corato, in visita dal gruppo Casillo, nel bel mezzo di una campagna elettorale, quali sono stati gli argomenti affrontati sul tema importazione grano estero? Quando si è recata da Casillo, *leader* del mercato dell'industria molitoria, lo ha invitato a dare precedenza e giusta valorizzazione al grano prodotto dagli agricoltori italiani da lei rappresentati? Dall'intervista questo non si evince. Con il suo messaggio, anziché promuovere l'utilizzo del grano italiano per la produzione di pasta e a tutela del *made in Italy*, ha invece ringraziato gli imprenditori industriali che effettuano la produzione di un *made in Italy* industriale ottenuto mediante la trasformazione di grano canadese. Il suo ruolo le impone di occuparsi della tutela del prodotto agricolo italiano, del grano italiano e non del prodotto industriale composto da materie prime canadesi.

il Ministero delle politiche agricole, che rappresento, è fortemente impegnato nel sostegno all'intera filiera cerealicola e in particolare a quella grano-pasta. A testimonianza di ciò, nel decreto rilancio ho fortemente voluto l'inserimento dell'esonero contributivo straordinario, previdenziale e assistenziale, per il periodo da gennaio a giugno 2020 anche per i cerealicoltori. Tale misura rappresenta uno dei principali strumenti di risposta che il Governo ha messo in campo in questa fase molto delicata per il Paese. Sul fronte della trasparenza, ricordo al senatore interrogante che proprio su iniziativa del Mipaaf è stato prorogato il decreto che rende obbligatoria l'origine in etichetta del grano utilizzato per la pasta, una scelta chiara per mettere il consumatore nelle condizioni di conoscere, in maniera consapevole e informata, gli alimenti che acquista. Sul fronte della formazione dei prezzi, come il senatore interrogante saprà, il Ministero ha aperto un confronto con la filiera per la costituzione di una commissione sperimentale nazionale per il prezzo indicativo. A causa della pandemia, il termine della raccolta delle deleghe per stabilire la rappresentanza del mondo produttivo in questa commissione è stata posticipata al 30 settembre. Ricordo, inoltre, che in queste settimane si è provveduto allo sblocco dei pagamenti degli aiuti al grano duro nazionale in contratti di filiera e sono in corso di pagamento, dal Ministero ad Agea, ulteriori 10 milioni di euro per la domanda 2019. Sono convinta che potenziare i contratti di filiera rappresenti una delle azioni strutturali più poderose al fine di valorizzare la qualità del grano nazionale e favorire la produzione di qualità di pasta al Sul fronte della vigilanza siamo tutti impegnati nella tutela massima del consumatore, come dimostrano le migliaia di controlli effettuati dagli organi preposti, sono consapevole della necessità di aiutare la produzione agricola nazionale di grano duro a produrre sempre più grano di qualità, tenuto conto che l'industria della pasta lo assorbe completamente e non siamo autosufficienti in questa produzione. Per quanto riguarda la richiesta di far riportare in fattura la dicitura «grano duro di importazione nazionalizzato» ricordo che sui documenti di tracciabilità dei lotti importati rimane l'indicazione che il grano è di origine estera. Riporto infine quanto segnalato dal Ministero della salute, rispetto ai controlli di loro competenza. I numerosi controlli sanitari, effettuati dai competenti uffici periferici, uffici periferici, operanti presso porti ed aeroporti italiani, non hanno riscontrato, da tre anni a questa parte, nessuna criticità riguardo alla presenza di glifosato sul grano di provenienza estera, che risulta conforme alla normativa sanitaria nazionale ed europea.

In Commissione abbiamo avuto modo di riferire ai funzionari dell'Icqrf che i dirigenti della Capitaneria di porto, in prevalenza Puglia e in

per i produttori in modo tale che non ci sia un legame stretto con il proprio organo di rappresentanza sindacale, perché gli agricoltori vorrebbero che questa attività fosse svolta in libertà e che quindi fosse garantita loro la piena possibilità di conferire questa delega a chiunque. Mi auguro che quanto prima la commissione venga istituita e convocata sia avviato un processo di armonizzazione delle quotazioni nazionali con il resto del mondo, dove i grani di scarsa qualità con residui tossicologici subiscono un declassamento

tema della criticità nel sistema assicurativo delle imprese agricole, che crediamo davvero importante per un settore, che, come il Ministro ha ricordato anche in precedenza, abbiamo evocato tanto in questi mesi e di cui abbiamo parlato tantissimo durante il *lockdown*.

l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 hanno messo in gravissima difficoltà le aziende del settore agroalimentare, con un calo di liquidità, che riguarda tutto il settore.

offre un sostegno economico alle imprese stesse, ma d'altra parte comporta anche un impegno economico per tali imprese, perché da qualche parte le risorse per stipulare le assicurazioni devono essere trovate. È vero che ci sono contributi nazionali e comunitari che comunitari che sono fondamentali e che in alcune situazioni possono diventare anche essenziali. Tali risorse sono davvero importanti. Come

per accelerare i pagamenti e sostenere, cercando di eliminare o limitare i rischi, questa filiera della vita, come anche lei l'ha chiamata poco fa, di cui tanto abbiamo parlato e che noi del Partito Democratico - come lei ben sa - crediamo

agricole alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevole senatrice, sono consapevole delle difficoltà in cui versa il mondo agricolo e della necessità di ottenere semplificazioni in tutte le procedure che riguardano l'intero settore. Molte iniziative sono state già intraprese, ma occorre continuare in tale direzione per agevolare quanto più possibile l'intero comparto. In tal senso, per semplificare la documentazione formale che accompagna i piani assicurativi individuali, è stata già avviata un'interlocuzione con la Commissione europea per verificare la possibilità di stabilire dei valori *standard* di resa o di valori, entro i quali l'agricoltore è esonerato dall'esibire documentazione per dimostrare i propri dati di resa aziendale. Per quanto riguarda poi l'accelerazione dei rimborsi assicurativi, segnalo che anche le misure assicurative agevolate si avvalgono delle semplificazioni previste dalle norme Covid. le erogazioni in agricoltura (Agea) della firma differita per il rilascio della documentazione, alla possibilità di pagare sotto condizione risolutiva, prima della presentazione della documentazione antimafia e, per gli aiuti nazionali, alla possibilità temporanea di procedere al pagamento senza la preventiva verifica di eventuali pendenze fiscali. Ulteriori semplificazioni sono state introdotte anche per i controlli *in loco* previsti a campione sulle domande presentate. Rilevo poi che l'incremento del numero di imprese agricole che usufruiscono dello strumento assicurativo rappresenta uno degli obiettivi della misura per la gestione dei rischi del programma di sviluppo rurale nazionale. Stiamo lavorando anche nell'ambito della prossima programmazione per far sì che questa opportunità venga utilizzata da tutte le imprese agricole, almeno per la copertura dei rischi catastrofali che periodicamente colpiscono i nostri territori agricoli e le loro economie. Accanto a questa misura verrà comunque mantenuto il sostegno anche agli altri strumenti, come le polizze a copertura dei rischi puntuali (come ad esempio la grandine), i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi. In ogni caso per un'adeguata gestione dei rischi da parte delle imprese agricole sarà necessario coordinare gli interventi con le Regioni che dovranno integrare gli strumenti presenti con misure di investimento preventive di assistenza tecnica e trasferimento di conoscenza. Queste ultime necessarie a creare una cultura imprenditoriale di gestione dei rischi. L'insieme dei provvedimenti dovrà garantire la resilienza delle imprese per l'adattamento ai cambiamenti climatici, ma anche eventi non previsti, ma prevedibili, come la crisi di mercato. Concludo confermando il mio massimo impegno a sostenere ogni iniziativa finalizzata all'adozione di misure di sostegno alle imprese del settore, che in questi ultimi mesi, nonostante le straordinarie difficoltà incontrate, hanno garantito la tenuta del sistema agricolo italiano.

che riguarda anche altre parti e altri piani del nostro tessuto aziendale nazionale: prendere il meglio da questa situazione di crisi per farlo diventare la normalità. Quello che lei dice sull'accelerazione dei rimborsi

e noi siamo a disposizione. Si è parlato tanto del rapporto tra Parlamento e Governo: noi siamo a sua completa disposizione per provare a dare una mano a un settore che ci sta tanto a cuore.

contenente tutta una serie di iniziative proprio per il turismo. Ciò sta a significare che ad oggi non è stato fatto molto, se non addirittura niente. Ci sono degli studi, molto autorevoli, che certificano che fino a maggio, a fronte dell'emergenza Covid, c'è stata una perdita netta di circa 275 miliardi. Dio non voglia che l'emergenza si allunghi fino a dicembre, perché in quel caso la stima la stima è di 640 miliardi. Provvedimento dopo provvedimento, dal cura Italia al liquidità e al rilancio, è evidente che le misure che sono state adottate non sono state sufficienti.

siccità. Siccome lei molto spesso ha fatto riferimento a risorse, provvedimenti, progetti e progettualità, noi siamo qua a chiederle - lo leggo, perché è importante che io legga bene quello che le chiediamo che le chiediamo - se siano già state individuate le risorse che verranno messe a disposizione del settore e gli interventi che il Governo intenderà realizzare attraverso la prossima manovra economica. Chiudo, signor Presidente, per stare all'interno dei tempi - come lei ci raccomanda - mostrando al Ministro un

senatore Centinaio, ha gestito il Ministero del turismo - come è capitato anche a me nell'altra legislatura - in un momento positivo di grande crescita e di sviluppo impetuoso, come è stato negli ultimi anni, del turismo internazionale in Italia. E capite bene, pur essendo all'opposizione oggi, che è completamente diverso gestire il Ministero non in una situazione di crescita, ma dentro un dramma enorme come quello che ha colpito il turismo in tutto il mondo dopo l'emergenza Covid. Sono state fatte molte cose nei provvedimenti. Non è un annuncio o un rinvio. Abbiamo fatto - mi dispiace doverle brevemente elencare - nei diversi decreti che si sono susseguiti l'esonero del versamento IRAP; il contributo a fondo perduto per il calo di fatturato; il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro; le agevolazioni per l'accesso alla liquidità; per la prima volta sono stati estesi al settore ammortizzatori sociali che il settore non ha mai avuto come la cassa integrazione in deroga

e i pacchetti turistici; il credito di imposta per le locazioni e l'affitto d'azienda; l'abolizione del versamento della prima rata IMU per il solo settore del turismo; il fondo per il turismo; il ristoro della tassa di soggiorno ai Comuni;

dover utilizzare questo termine che - immagino - verrà criticato. Io non ho l'abitudine di venire in Parlamento ad annunciare dei provvedimenti prima che vengano discussi e approvati in Consiglio dei ministri. Posso dire su cosa stiamo lavorando perché è questione di giorni. Avremo due tappe importanti: una riguarda il decreto che faremo all'inizio di agosto, con le risorse

stiamo lavorando su tre priorità: la prima è garantire un sistema di ammortizzatori sociali per i settori che hanno crisi prolungate e, quindi, soprattutto il turismo (prolungamento della cassa integrazione e dell'indennità straordinaria per i lavoratori stagionali atipici); sostegno alle imprese, compreso l'IMU

in particolare per le agenzie di viaggi e i *tour operator*, che non hanno più clientela perché nessuno programma viaggi nel lungo termine e, quindi, hanno bisogno di un sostegno ben più forte dei primi 25 milioni che hanno già avuto. Il secondo settore è quello delle città d'arte perché, se il turismo è ripreso in alcuni settori, nelle città d'arte, purtroppo, c'è un problema particolare che richiede interventi ulteriori. Penso che il senatore Centinaio replicherà dicendo che sono insufficienti e inadeguati. Io volevo dirvi - lo ripeto - che continuerò a prendere ogni critica, anche la più ingenerosa, come un contributo positivo.

decreto-legge rilancio che l'indifferenza manifestata nei confronti del settore non è più accettabile. L'11 luglio, Federalberghi ha detto che a giugno c'è stato il meno 80 per cento. Il 27 luglio, Federturismo:

che il ministro Franceschini sta lavorando bene, noi saremo al fianco del ministro Franceschini. In caso contrario, la bocciamo, come la sta bocciando ora tutto il settore.

*(M5S)*. Signor Ministro, lo scorso 22 aprile, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, nominata il 14 maggio 2019, ha presentato in videoconferenza il nuovo logo del monumento vanvitelliano preannunciando anche e in che modo si intendesse riorganizzare il sito museale per il dopo Covid-19. A poche ore dal lancio del nuovo *brand* Reggia di Caserta, sui *social* sono comparsi commenti esclusivamente negativi. In particolare, il presidente dell'ordine degli architetti di Caserta Raffaele Cecoro ha affermato che che presenta una stretta connessione con la cultura e con il design, per questo motivo sento l'obbligo di dissentire in maniera molto forte per la scelta del nuovo logo della Reggia di Caserta. Caserta' manca totalmente di ogni riferimento storico-artistico e sembra un vero e proprio plagio in quanto simile se non identico ad altri loghi già esistenti. Sembra essere stato preso in prestito da quello del celebre campione di tennis Roger Federer da quello della nota società immobiliare canadese 'Ricco Colinares' che utilizza questo marchio da anni"; il lavoro per realizzare il *logo* "Reggia di Caserta" è stato assegnato con affidamento diretto, ai sensi con sede a Levata di Curtatone (Mantova), per l'importo di 37.500 al netto di IVA, autorizzato dall'allora direttore *ad interim* Antonio Lampis. L'agenzia Sigla Comunicazione di Mantova ha prodotto un logo estremamente semplice, che non lascia intravedere alcuno sforzo creativo sia grafico che storico, con l'uso banale delle iniziali «R» e «C». Considerato che il nuovo logo della Reggia di Caserta non rappresenta i caratteri profondi che connotano il monumento, la semplicità grafica ha dato adito alla profusione di numerose parodie, tanto da far temere un danno di immagine al monumento stesso. Inoltre, è parere degli interroganti che la paventata aria di cambiamento che si vuole promuovere per la Reggia di Caserta non si addica in alcun modo al prestigio del monumento, che si ricorda essere patrimonio Unesco ed uno dei più visitati d'Italia. Peraltro, il logo preesistente, che raffigurava la piantina della Reggia di Caserta vista dall'alto, a detta di tutti era molto più rappresentativo. Considerato, infine, che il costo per la realizzazione del nuovo logo è stato di 37.500 euro, cifra significativa, soprattutto in considerazione del periodo di crisi che detta cifra poteva essere utilizzata per interventi mirati di riqualificazione e manutenzione dei parchi e degli edifici, si chiede di sapere quanto l'iniziativa descritta abbia causato un danno di immagine ed economico non solo alla Reggia di Caserta, ma anche all'intero patrimonio culturale italiano, e soprattutto quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere per porre rimedio a quello che potremmo considerare un vero e proprio oltraggio alla storia.

i direttori dei più grandi musei italiani, ha portato una ventata di innovazione: restauri, riqualificazione del parco, aumento del numero dei visitatori, miglioramento dei servizi riconosciuto in modo assolutamente trasversale e, soprattutto, fuori dai confini del nostro Paese, visto anche l'enorme aumento del numero dei visitatori. In conseguenza di questo lavoro di rinnovamento, nel 2019 il direttore museale *ad interim* *ad interim* - il direttore precedente, Felicori, era andato in pensione - ha ravvisato la necessità di riorganizzare il sito e di cercare un *brand*, un logo che lo promuovesse in modo più efficace. È stata avviata

È naturale che vi sia un dibattito quando si introduce un logo nuovo, ma è stata largamente prevalente la valutazione negativa. Il *brand* Reggia di Caserta come logo tipo adesso è oggetto di una valutazione: non ci Il nuovo direttore della Reggia di Caserta ha deciso di promuovere, e sta già facendo, un concorso internazionale per la scelta del logo. quindi, che tutto questo potrà essere tranquillamente superato. Aggiungo - lo dico perché, essendo stata presentata un'interrogazione, ovviamente ho il dovere di rispondere - che, rispetto al rapporto tra istituzioni museali e politica,

autonoma dei musei e quindi le scelte, positive o negative, debbano restare nella totale autonomia. Pertanto, né noi come politici, né tantomeno io come Ministro, possiamo metterci a valutare la singola scelta, giudicandola, anche in base a criteri molto soggettivi, molto soggettivi, giusta o sbagliata, quando soprattutto riguarda le politiche di comunicazione di un museo. Detto questo, mi pare che la spinta dell'opinione pubblica abbia portato a rivedere la scelta da parte della direzione

possa creare un po' di difficoltà di affiliazione, di amorevole affetto nei confronti di un metodo di gestione rispetto al rapporto reale che ci dovrebbe essere tra una città e il territorio. Siamo rimasti già colpiti dal fatto che sono bastati dieci giorni per fare un passo indietro da parte della direttrice: in realtà, già in un comunicato stampa del 29 aprile si diceva che il logo in parte veniva ritirato. Sono andata personalmente alla Reggia

utilizzato ad ora è scomparso l'ologramma della piccola corona e non ci sono i famosi quattro cortili, che erano stati molto ben accetti non ma anche dal mondo della cultura italiano, in quanto, con un semplice segno grafico, essi rappresentavano perfettamente la Reggia di Caserta. Ci siamo informati anche noi sull'eventualità di voler procedere quanto prima con un concorso internazionale di idee e ci auguriamo che, anche da parte sua, ci sia una sollecitazione perché questo avvenga presto, perché credo che la Reggia meriti una particolare attenzione.

UV))*. Signor Ministro, come sappiamo, l'Italia ha subordinato l'ingresso dall'estero all'andamento della curva dei contagi nei Paesi di provenienza. Da alcuni è stata completamente ripristinata la libera circolazione; da altri, tra cui anche i Paesi europei come la Bulgaria e la Romania, è stato introdotto l'obbligo di quarantena. Da altri ancora non vi è la possibilità di accedere in Italia, se non per comprovati motivi di lavoro di studio di salute. Tra questi ce ne sono diversi che hanno fitte relazioni con l'Italia: il Bangladesh, il Brasile, la Macedonia del Nord, la Bosnia-Erzegovina, solo per citarne alcuni. La questione interessa madri e padri separati dai loro figli, ma anche coppie, sposate o meno, che hanno il diritto di ricongiungersi con la persona con la quale hanno un legame sentimentale stabile. Queste persone, che si sono associate in una rete di nome "Love is not tourism", hanno dichiarato la loro disponibilità a effettuare, eventualmente anche a loro spese, i necessari test, sia all'arrivo sia alla partenza, con controlli periodici, anche settimanali. Inoltre, a quanto risulta, i Governi di Danimarca, Norvegia e Olanda hanno già provveduto ad inserire questi soggetti tra quelli esenti dal divieto di transito. Tutto ciò premesso, si chiede di sapere se il Ministro non ritenga opportuno prendere provvedimenti affinché anche in Italia i soggetti interessati e rientranti nella categoria siano inseriti

di fare un punto su una vicenda assolutamente rilevante. Negli ultimi mesi siamo riusciti a piegare la curva del contagio, tra mille difficoltà che sono note, chiaramente, agli onorevoli senatori presenti, grazie soprattutto ai comportamenti virtuosi delle italiane e degli italiani e grazie a misure molto dure assunte dal Governo nazionale e dalle nostre Regioni. Ho già avuto modo di dire in quest'Aula che siamo fuori dalla tempesta, ma non siamo ancora in un porto sicuro. Intanto, la situazione internazionale, quella al di fuori dei confini del nostro Paese, è purtroppo sempre più complicata. Siamo arrivati ad oltre 17 milioni di casi, con oltre un milione di casi in più a settimana e, purtroppo, una situazione neanche sotto controllo nella nostra Europa, in modo particolare nei Balcani. Ahimè, però, negli ultimi giorni ci sono segnali non positivi che vengono anche da importantissimi Paesi europei quali la Francia, la Spagna e la Germania. Dentro questo contesto, sono stato costretto, per difendere il nostro Paese, a firmare ordinanze molto stringenti, non solo per tutti i Paesi extraeuropei ed extra-Schengen con l'obbligo di quarantena, ma anche nei confronti due Paesi europei come Romania e Bulgaria, che sono costretti alle stesse misure dei Paesi extraeuropei. Queste sono scelte dolorose, che nessuno di noi fa a cuor leggero, ma sono scelte indispensabili per difendere il nostro Paese e per non vanificare i sacrifici enormi che le italiane e gli italiani hanno compiuto finora. Sulla base di queste valutazioni, voglio dirle che valuterò con la massima attenzione le sue riflessioni e proposte, perché toccano un tema che mi sta particolarmente a cuore e che ha a che fare con diritti di natura costituzionale, riconosciuti nel nostro Paese come quelli che tutelano le relazioni di natura familiare. Valuterò, quindi, con la massima attenzione

tumori piuttosto che malattie cardiovascolari o altro. In questo senso, l'allungamento delle liste di attesa comporta un gravissimo problema per la popolazione italiana proprio per i livelli di assistenza che possiamo garantire ai cittadini italiani. Sa benissimo che c'è una situazione frammentaria, Ministro, e con la nostra interrogazione le chiediamo innanzi tutto di conoscere la situazione Regione per Regione, perché abbiamo notizie molto varie; quindi, un intervento nazionale, che ovviamente deve portare avanti il Governo per evitare disuguaglianze esistenti certamente a livello territoriale e non

ha detto bene: non vi è dubbio che negli ultimi mesi il Servizio sanitario nazionale abbia impegnato tutte le proprie energie per affrontare l'emergenza Covid e non poteva oggettivamente che essere così. I nostri medici e infermieri hanno incessantemente usato tutte le ore a loro disposizione per fronteggiare

di ricominciare a occuparci di tutte le funzioni ordinarie del Servizio sanitario nazionale, perché c'è una grande verità: il Covid è stato il nostro primo nemico degli ultimi mesi, ma non ha fermato le altre patologie

Noi siamo al lavoro su questo punto attraverso due gambe sostanziali: la prima è una ricognizione puntuale, che stiamo facendo già da alcuni giorni, in collaborazione con tutte le Regioni, per capire qual è il fabbisogno esatto di cui stiamo parlando; la seconda dovrà essere la messa in campo, immediatamente, di nuove risorse per un vero e proprio piano straordinario di nuovi investimenti per recuperare le liste di attesa. Posso dire sin da oggi che nel prossimo decreto che si adotterà all'inizio di agosto, per effetto dello scostamento che proprio ieri il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati hanno autorizzato, indicheremo risorse molto significative che io ho chiesto al Ministro dell'economia proprio per finanziare questo piano straordinario. Voglio dire che il Servizio sanitario nazionale non si fermerà in estate: proveremo ad allargare orari e giorni di disponibilità per rispondere a questa esigenza. Abbiamo chiaramente bisogno di più risorse. Mi permetta qui solo di ricordare che negli ultimi cinque mesi sul Servizio sanitario nazionale sono state messe più risorse che negli ultimi cinque anni; non c'era mai stato nella storia di questo Paese un investimento così forte. *(Applausi)*. Io penso che sia la strada giusta e lavoreremo da subito per rispondere a questa esigenza.

siamo molto preoccupati per quello che può avvenire da qui ai prossimi mesi, perché il problema delle lunghe liste di attesa esiste

avanzato delle proposte, mai in maniera scomposta, ma sempre nella direzione dell'interesse della nostra Nazione e del nostro popolo. Noi vogliamo veramente che venga fatto

grazie, c'è stata la pandemia e volevo vedere se non riuscivamo a fare questo. Dobbiamo fare ancora di più e molto meglio, perché le liste di attesa in un Paese civile a livello mondiale come l'Italia non possono essere accettate perché sono proprie di

**Interrogazione sull'interruzione delle prestazioni sanitarie destinate ai minori con disabilità** Ministro, come lei sa bene, noi siamo intervenuti più volte a tutela dei diritti dei bambini portatori di *handicap* e, quindi, a sostegno delle loro famiglie.

di difficoltà più specificamente di tipo motorio o anche a quelli considerati portatori di disagio sul piano delle competenze di tipo cognitivo, di cui spesso ignoriamo le ragioni del ritardo, che però sono reali e che definiscono questo piccolo universo di bambini portatori di *handicap.* Ebbene, questi bambini sono stati i più penalizzati in occasione del recente *lockdown*, e lo sono stati per una ragione molto semplice: prima di tutto non hanno ricevuto quel tipo di supporto specifico che i centri specializzati offrono loro.

in modo particolare questo lavoro tocca sempre alle madri, che hanno svolto nei loro confronti ogni tipo di attività possibile. La cosa peggiore è che, mentre si sono riaperte mille altre strutture mille altre strutture - ovviamente sappiamo bene che non si è riaperta la scuola - non si sono riaperti neppure i centri altamente specializzati che si occupano di questi bambini e che avrebbero perfettamente potuto attrezzarsi per la loro accoglienza.

il secondo è la possibilità che vengano reintegrati i periodi di mancato sostegno attraverso forme di supporto personale e il terzo - quello che mi preoccupa altrettanto e probabilmente più - è che lei si faccia interprete presso la sua collega Ministro dell'istruzione perché a questi bambini non manchi nulla, nemmeno l'opportunità di un solo giorno in cui possano andare a scuola e ricevere tutto l'aiuto di cui hanno bisogno.

che tocca tutte le nostre coscienze. Io ho letto con molta attenzione la sua interrogazione, che considero densa di spunti interessanti per il lavoro delle prossime settimane. Da parte mia c'è tutta la volontà di dare risposta positiva a tutte e tre le questioni che lei ha provato a porre. Io sono d'accordo su un punto di fondo, che credo valga in modo particolare per i nostri bambini più fragili in situazioni di difficoltà, ma forse anche più in generale per tutte le fragilità del nostro Paese. Non vi è alcun dubbio che tutto il Paese abbia pagato un prezzo enorme per il *lockdown,* ma ha pagato un prezzo ancora più alto chi era in una situazione di maggiore debolezza. In sostanza, che il *lockdown* ha provocato un aumento delle diseguaglianze, perché chi è più forte naturalmente riesce ad affrontare meglio una situazione nuova, molto complicata e molto difficile. E penso che questo sia un tema di cui dobbiamo necessariamente occuparci. come farlo, io credo che ci sia bisogno di un ruolo forte e nuovo dello Stato e in modo particolare dell'apertura di una nuova stagione di investimenti. Non voglio tornare sempre su questo punto, ma ritengo che la questione essenziale sia sempre la seguente: veniamo da una stagione troppo lunga, nella quale al Servizio sanitario nazionale sono stati operati tagli irricevibili e dobbiamo avere il coraggio di dire che quella stagione dei tagli è definitivamente chiusa e che si apre, invece, una nuova, grande stagione di investimenti. Abbiamo iniziato a farlo, non basta, ma questa è la direzione giusta. Penso, ad esempio, al decreto rilancio, ai 750 milioni di euro che abbiamo stanziato per l'assistenza domiciliare, che è un grande intervento che prova a rispondere ad almeno una parte delle fragilità che anche lei ha velocemente indicato. Infine, mi consenta di ricordare un punto, che era contenuto nell'interrogazione e che a me sembra di particolare rilievo. Nella giornata del 28 luglio ho istituito la nuova Commissione per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Credo che lì si giochi una partita strategica per il nostro Paese. I livelli essenziali di assistenza sono i servizi fondamentali che il nostro Stato gratuitamente offre ad ogni persona e rappresentano il simbolo più bello dell'articolo dell'articolo 32 della nostra Costituzione, che dobbiamo difendere con tutta l'energia che abbiamo, rimettendo al centro sempre quel cittadino-paziente che io credo debba essere il vero cuore del nostro Servizio sanitario nazionale.

credendo davvero che ci sia l'intenzione di supplire alle carenze che si presenteranno nella situazione che stiamo per vivere, ma anche con la consapevolezza che abbiamo mancato di assumerci le responsabilità per i fatti che sono appena accaduti. C'è un desiderio quasi risarcitorio nei confronti di questi bambini e delle loro famiglie, che richiede da parte nostra un impegno rinnovato. Ministro, un aspetto mi sembra particolarmente importante. Ci troviamo davanti a bambini in età evolutiva e stiamo difendendo i loro diritti. Il fatto che oggi ci carichiamo del loro diritto alla del loro diritto alla salute, ma anche a ricevere tutti i mezzi necessari per raggiungere la massima autonomia possibile all'interno della loro situazione, significa per lei

Il diritto alla salute non è un costo: tutelarlo è un investimento e, se si tratta di minori con difficoltà, è un dovere morale per tutti noi.

si procederà allo scrutinio e alla proclamazione del risultato. Se qualcuno deve votare, può farlo passando sotto i banchi della Presidenza.

dei voti. Proclamo pertanto il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Matteo Salvini, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* (Doc. IV-*bis*, n. 3): |

Allegato B).* Ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento, a causa del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, le conclusioni

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della prossima settimana. La giornata di martedì 4 agosto sarà dedicata ai lavori delle Commissioni. L'Assemblea si riunirà nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 per discutere i seguenti argomenti: il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione con l'Argentina nel settore della difesa; la relazione della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti relativa all'emergenza epidemiologica Covid-19. Alle ore 15 di giovedì 6 agosto avrà luogo il *question time*.

Signor Presidente, porto in Aula la protesta di centinaia di migliaia di cittadini dell'Abruzzo, del Lazio e della Campania, alle prese con il disastro provocato dall'inquinamento del fiume Liri, da decenni oggetto, da un lato di sfruttamento e sversamenti incondizionati, dall'altro di difesa e tutela da parte di associazioni e cittadini. Tra le problematiche, il massiccio sfruttamento da parte delle centrali idroelettriche - ben sei - nonché una serie di episodi che hanno evidenziato fenomeni di schiuma, inquinamento e moria di pesci. Per quanto riguarda lo sfruttamento idroelettrico, una politica dissennata e brutale ha portato settant'anni fa addirittura alla deviazione del fiume all'interno di una galleria scavata nei Monti Simbruini per poter alimentare a valle delle centrali idroelettriche. Questa scelta scellerata ha portato all'annientamento di un'economia e di una cultura millenaria legata al fiume, alle sue risorse e alle sue attività economiche, peraltro scatenando un impoverimento così drammatico da provocare una migrazione di massa e lo spopolamento di interi paesi, a cominciare da Castellafiume, che ancora oggi scontano questa privazione. Per tutto ciò chiedo che il fiume sia restituito al suo corso millenario per ridare almeno fiato alle iniziative ambientali e turistiche che si potrebbero in breve tempo avviare. poi l'altro aspetto dell'incuria; già nel settembre 2017 a Civitella Roveto era stata rilevata acqua di un colore violaceo. A seguito di questo episodio numerose associazioni si sono costituite sul territorio, associazioni che oggi denunciano sfruttamento e inquinamento del fiume, come è accaduto nel mese di maggio a seguito di una misteriosa schiuma rilevata all'altezza del Comune di Capistrello e dell'emissario che nel fiume fa confluire confluire le acque proveniente dalla Piana del Fucino. L'allarme è scattato; ci sono state riunioni con i sindaci, il Consorzio acquedottistico marsicano, la cartiera Grazie a tutti Degli impianti di depurazione dei Comuni da più fonti definiti non in regola? Siamo in attesa di sapere e conoscere. Nel frattempo, chiedo al ministro dell'ambiente Costa di intervenire per valutare la portata del disastro e all'Enel e agli altri enti coinvolti di valutare immediatamente la possibilità di cancellare la vergogna della deviazione del fiume per alimentare centrali elettriche, che oggi potrebbero essere sostituite da altre Nel frattempo, chiedo al ministro dell'ambiente Costa di intervenire per valutare la portata del disastro e all'Enel e agli altri enti coinvolti di valutare immediatamente la possibilità di cancellare la vergogna della deviazione del fiume per alimentare centrali elettriche, che oggi potrebbero essere sostituite da altre fonti di produzione